L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legge di contabilità e finanza pubblica ha delineato un nuovo processo di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, della ripartizione degli stessi tra i sottosettori della pubblica amministrazione, nonché delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Ricordo in proposito che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, la Decisione di finanza pubblica (la cosiddetta deve esporre anzitutto, almeno per il triennio successivo, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, le previsioni tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa e del debito, sia complessivi che articolati per i sottosettori istituzionali, e gli obiettivi programmatici dei saldi e del debito per il complesso delle amministrazioni pubbliche e per i suoi sottosettori, al netto e al lordo degli interessi e delle misure *una tantum*, espressi in percentuale del prodotto interno lordo. Nel delineare gli scenari economici in atto, il documento in esame riferisce anzitutto che nel primo semestre del 2010 l'economia mondiale ha continuato a crescere a un ritmo sostenuto, così come il commercio mondiale. L'inflazione è rimasta sotto controllo anche in virtù dell'elevato grado di capacità produttiva inutilizzata generato dalla crisi. Nell'area dell'euro, in particolare, il PIL è cresciuto, in termini congiunturali, dell'1 per cento. I contributi maggiori sono venuti dai consumi privati (0,3 punti percentuali) e dagli investimenti fissi (sempre 0,3 punti percentuali). Questo risultato fa seguito a una crescita del PIL nel primo trimestre pari allo 0,3 per cento sul trimestre precedente, a cui aveva principalmente contribuito l'aumento delle scorte, per 0,8 punti percentuali. Tra i diversi Paesi dell'area, il documento sottolinea che la ripresa è però risultata differenziata, sia nell'entità sia nelle principali determinanti della crescita del PIL, alcuni Paesi hanno mostrato difficoltà nel cogliere appieno l'opportunità di risalire nel ciclo. Per l'Italia, in particolare, i dati sembrano mostrare un certo consolidamento della ripresa iniziata agli inizi dell'anno. Pur con l'incertezza che ancora caratterizza l'economia internazionale (in questi giorni l'OCSE ha diramato il suo «superindice» che indica un prossimo rallentamento nella crescita dei principali Paesi)

Così come per il mercato del lavoro, l'occupazione nel secondo trimestre, seppure in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (con una diminuzione dello 0,8 per cento), segna un confortante aumento

un tema, quello dell'occupazione, che riveste un posto sempre più rilevante nella discussione politica, culturale e anche accademica, non solo domestica. Non è un caso che il Premio Nobel per l'economia sia stato assegnato quest'anno a tre autorevoli studiosi che hanno indagato le difficoltà

Tuttavia, su quei due riferimenti appena accennati è forse necessaria qualche riflessione: seppure significativi, non riescono a dare il senso della complessiva situazione economica nazionale. Essi infatti andrebbero letti e valutati insieme ad altre informazioni - per così dire "macro" - dell'economia reale, rapportando il tutto alla situazione degli altri Paesi protagonisti in questi anni sulla scena dell'economia globalizzata: l'andamento del PIL, che dovrebbe fare i conti con un'economia che pesa sensibilmente e più che in altri Paesi; l'*export*, ovvero uno dei due pilastri su cui dovrà basarsi il rilancio del nostro Paese e che nel primo semestre di quest'anno ha dato segnali di chiara ripresa. Anche dall'ultimo dato ufficiale (quello di agosto) emergono - come si legge nel comunicato dell'ISTAT - incrementi tendenziali delle esportazioni verso tutti i principali partner commerciali, comunitari certo, ma soprattutto *extra* UE, come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia e il Brasile. Sono dati inferiori solo a quelli realizzati dalla Germania e portano il nostro Paese dietro a Germania e Gran Bretagna nella classifica della propensione all'*export*. andamento positivo ha interessato diversi settori, da quello energetico a quello dei macchinari, dal tessile dell'abbigliamento alle materie plastiche: segnale che la struttura industriale italiana conserva la capacità di reggere in questa difficile fase post-crisi, forse anche perché in corso una significativa ristrutturazione dell'apparato produttivo. Tali cambiamenti stanno segnando profondamente un Paese in cui non ci sono più politiche di svalutazione e vincoli alla libera circolazione di merci, capitali e persone. Un Paese che sta mutando struttura industriale: i suoi picchi stanno lasciando il posto alle piccole colline - come ha detto qualcuno - dalle quali, però, non è impossibile guardare lontano. I prezzi in qualche modo vanno raffreddandosi: l'indice dei prezzi al minuto, che a luglio aveva segnato un più 1,7 rispetto allo stesso mese del 2009, ad agosto è sceso a più 1,6.

Gli stipendi e le retribuzioni, certamente inferiori a quelli di partner come la Germania, nel primo semestre di quest'anno hanno fatto registrare una crescita significativa (soprattutto nel settore privato), superiore a quella dell'inflazione, che continua ad attestarsi oltre il 2 per cento rispetto all'agosto del 2009, dell'*annus horribilis*. in sintesi, di una situazione che non vuole nascondere le difficoltà e le incertezze che ancora gravano sulla nostra economia e non vuole nascondere quanto è necessario fare sul fronte delle infrastrutture della gestione del debito, per agganciare la possibile ripresa ed innestare un crescita robusta. Essa vuole soltanto invitare ad una riflessione su quale sia il reale contesto economico; una riflessione svolta in maniera non ideologica, come nel caso del declinismo a tutti i costi che da tempo ormai pervade la comunicazione, che dovrebbe portare invece ad un sereno approfondimento che consenta di individuare rigorose politiche procicliche. Nondimeno, secondo il documento, il 2010 dovrebbe registrare a consuntivo una revisione al rialzo della crescita di 0,2 punti percentuali, all'1,2 per cento, e una revisione al ribasso di pari entità, che dovrebbe riflettersi solo nel 2011, all'1,3 per cento, rispetto ai dati contenuti nella RUEF della scorsa primavera. Nel biennio 2012-2013, la crescita del PIL si attesterebbe così al 2 per cento in ciascun anno, andando a ridurre in parte l'ancor ampio *gap* di capacità produttiva inutilizzata. Quanto agli andamenti tendenziali riferibili ai saldi di finanza pubblica, il documento specifica che lo scenario considerato sconta tutti gli effetti del decreto-legge n. 78 del 31 con il quale il Governo ha ritenuto di dover anticipare all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013, e conferma gli obiettivi indicati nella RUEF. Il documento stima l'incidenza del debito sul prodotto, che dovrebbe salire di circa 2,5 punti, al 118,5 per cento del PIL, e il disavanzo, per il 2010, al 5 per cento dello stesso PIL. Un dato, quest'ultimo, certamente raggiungibile, considerando l'andamento del quadro complessivo, che costituisce un segnale di riequilibrio dei conti pubblici, premessa necessaria per un più robusto rilancio dell'economia. Un dato, poi, che insieme al deficit della Germania è tra i migliori tra quelli stimati dal Fondo monetario internazionale per il 2010. Le stime indicano un profilo di riduzione del disavanzo nel triennio 2011-2013, in coerenza con quanto indicato nel Programma di stabilità presentato all'Unione europea all'inizio dell'anno. In particolare, con la manovra di luglio il saldo di bilancio tendenziale è stato ridotto di un ammontare pari a circa 12 miliardi nel 2011 e a circa 25 miliardi in ciascuno dei due esercizi successivi, a fronte di una manovra lorda (sotto forma di maggiori entrate e di minori spese) pari, complessivamente, a 17,8 miliardi nel 2011, 27,5 miliardi nel 2012 La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento del PIL, dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dal riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS e alle entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale-*ter*), viene indicata nei dati di previsione in costante riduzione, attestandosi a fine periodo 2013, al 42,4 per Nello specifico degli andamenti previsti, il dato relativo all'andamento delle entrate complessive dovrebbe risentire del ridursi progressivamente della loro incidenza rispetto al PIL nel triennio (dal 47,2 per cento del 2009 al 46,4 per cento del 2013), a causa della riduzione sia dei contributi sociali che delle entrate tributarie. Per quanto concerne in particolare le entrate tributarie, esse sono previste in riduzione al 28,8 per cento rispetto al PIL del 2010, dal 29,1 per cento del 2009, e rimangono sostanzialmente stabili sino al 2013, per cui la flessione del 2010 sarebbe da ascriversi all'inclusione nel 2009 di entrate *una tantum*, pari allo 0,8 per cento del PIL (dovute al recente scudo fiscale e all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze), tanto che, al netto di tali introiti, dette entrate presenterebbero una crescita, lieve lieve e circoscritta, dello 0,5 per cento rispetto al PIL. Quanto ai dati della spesa, il loro valore totale al netto degli interessi, in rapporto al PIL, evidenzia nello scenario riportato dal documento una significativa riduzione (meno 4 punti percentuali di PIL),

La spesa totale presenta, nel periodo 2010-2013, un tasso di crescita cumulato pari al 5,3 per cento; al netto degli oneri per interessi, l'incremento si riduce al 3,7 Se si prende in riferimento il triennio 2011-2013, il tasso di crescita della spesa è pari al 4,2 per cento, e si riduce al 3 al netto degli interessi. Tale dinamica evolutiva, inferiore a quella prevista per il PIL, determina una riduzione della spesa al netto degli interessi di 3,5 punti percentuali di PIL, passando dal 47,3 del 2010 al 43,8 per cento

Le spese in conto capitale presentano nel triennio di previsione una riduzione rispetto al PIL (meno 1,3 punti percentuali di PIL), molto più contenuta di quella stimata per le spese correnti al netto degli interessi (meno 2,7 punti percentuali di PIL), anche per effetto di politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica. Il documento reca inoltre una specifica trattazione relativa al tema del debito pubblico. Negli andamenti attesi, il debito pubblico inizierebbe a ridursi a partire dal 2012, raggiungendo il 115,2 per cento nell'anno successivo. L'andamento del rapporto debito/PIL che ne consegue per gli anni 2009-2012, già precedentemente evidenziato, conferma sostanzialmente quanto previsto nella Il documento sottolinea peraltro come una parte significativa della dinamica del debito della pubblica amministrazione sia dovuta alle amministrazioni centrali (il cui debito passa da 1.659 miliardi di euro del 2009 a 1.886 miliardi nel 2013), mentre il debito delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza rimane di fatto stabile nell'arco di tempo considerato. Quanto invece alla spesa per interessi, connessa al debito, le stime riportate nel documento prevedono una riduzione significativa rispetto alla RUEF per gli anni 2011 e 2012, spiegata in larga parte con la riduzione dei tassi, rispettivamente dello 0,2 e dello 0,4 per cento. Nel complesso, l'impostazione del documento risulta coerente con il quadro di rafforzamento delle procedure di controllo della qualità dei dati di finanza pubblica delineato in ambito europeo con il nuovo pacchetto di proposte normative approvato dalla Commissione lo scorso 29 settembre. In tal senso, la riforma ancora in via di completa definizione della *governance* europea segna un passaggio importante per definire un meccanismo efficace per la gestione delle crisi, anche predisponendo procedure chiare e credibili per la concessione tempestiva di assistenza agli Stati membri in serie difficoltà finanziarie. di vista, gli indirizzi assunti dalla Commissione europea sembrano proporre una correzione del Patto di stabilità e crescita che preveda, assieme ad un più stretto coordinamento *ex ante* delle politiche di bilancio, un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori e una maggiore enfasi sugli obiettivi di debito e sulla sostenibilità dei conti pubblici. Difatti, nell'ambito del progetto di riforma presentato alla fine di settembre, la Commissione propone di rendere operativa la regola della procedura per i disavanzi eccessivi relativa al debito, in base alla quale l'incidenza sul PIL del debito delle amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al 60 per cento e, se superiore, deve diminuire ad un ritmo adeguato. Presidente, colleghi, sintetizzando l'azione di politica economica delineata nella Decisione di finanza pubblica, va rilevato come l'ineludibile azione di contenimento del livello dell'indebitamento sia prevalentemente prefigurata attraverso un significativo ridimensionamento delle uscite complessive, pari a circa 26 miliardi nel periodo 2011-2013, conseguente alle rigorose politiche di riqualificazione della spesa pubblica e di riduzione delle spese improduttive perseguite dal Governo durante tutto l'arco della legislatura. Ci conforta il fatto che, nonostante gli effetti negativi determinati anche sotto questo profilo dalla recessione economica, le entrate tributarie mostrino una sostanziale tenuta lungo l'arco temporale considerato dalla Decisione di finanza pubblica, in quanto la tendenziale riduzione del gettito delle imposte dirette dovrebbe essere bilanciata dal miglioramento nell'andamento delle imposte indirette. In tale contesto, è evidente la necessità di proseguire, a livello nazionale, in un'impostazione di politica economica che coniughi l'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con quella di liberare il più possibile risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali. Nella medesima prospettiva, è altrettanto necessario avviare un processo di revisione e semplificazione del sistema tributario, che consenta di perseguire l'obiettivo programmatico della progressiva riduzione della pressione fiscale, in un quadro di piena responsabilità di bilancio. A margine, rilevo anche l'esigenza di evitare che l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea 3, volto a rafforzare i meccanismi per garantire l'adeguatezza patrimoniale delle banche a fronte dei finanziamenti da loro erogati, non determini effetti negativi sull'effettiva disponibilità di credito per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese. A conclusione di queste brevi note, sottolineo la necessità che la discussione in sede UE sulle proposte legislative di riforma sia affrontata dal Governo, nonché da tutte le componenti politiche ed istituzionali del Paese, con la massima attenzione e consapevolezza, trattandosi di un passaggio cruciale che condizionerà le prospettive, economiche e politiche, della stessa Unione ed inciderà fortemente sulle opzioni di politica economica di lungo periodo di ciascuno degli Stati membri. *(Applausi finestra"). Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale per geometri «Enrico Fermi» di Lanciano, in provincia di Chieti. A loro rivolgiamo

minoranza*. Signor Presidente, colleghi, sostiene il Governo, in premessa alla Decisione di finanza pubblica che, cito testualmente, «questo documento è sostanzialmente e politicamente superato». Non solo perché solo perché «quanto doveva essere deciso è già stato deciso a luglio», ma soprattutto perché i «nuovi documenti contabili europei (...) avranno da subito una loro propria centralità politica, assoluta e assorbente». Di qui la scelta politica di negare rilievo alla Decisione di finanza pubblica al nostro esame. È una scelta politica che noi non condividiamo. Anzi, è una scelta politica che noi radicalmente avversiamo: non perché vogliamo negare la centralità delle decisioni e delle scelte che si prenderanno nel corso della prossima sessione di bilancio europea, ma esattamente per la ragione opposta. Colleghi, entro il 12 novembre prossimo, cioè tra un mese, l'Italia dovrà presentare alle istituzioni comunitarie la versione preliminare del Piano nazionale di riforma elaborato nell'ambito della nuova Strategia dell'Unione 2020. Questa versione preliminare del piano nazionale di riforma dovrà essere predisposta tenendo conto dello scenario macroeconomico a medio termine e dovrà concentrarsi,

Dovrà identificare gli ostacoli principali che si oppongono al conseguimento degli stessi obiettivi di crescita e di aumento dell'occupazione, definendo le misure che il Paese intende adottare per superarli. Allora, colleghi, mettiamo un po' in ordine date, scadenze e relative scelte politiche. Se per il 12 novembre, cioè tra un mese, il Governo deve portare in Europa la versione preliminare di questo Piano, come non considerare preziosa l'occasione rappresentata, per un'adeguata preparazione di una scelta tanto impegnativa, dalla discussione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica? Ricordo che con la votazione di una risoluzione parlamentare che potrebbe e dovrebbe essere l'atto di indirizzo rivolto al Governo per la predisposizione della bozza di Piano nazionale di riforma?

La risposta burocratica - del Governo (se capisco, supinamente accettata da tutte le forze della maggioranza) non trova dunque alcun fondamento nella prossima "sessione di bilancio" europea. La scelta del Governo - rinviare il confronto sulle scelte impegnative e difficili alla prossima primavera, derubricando a carta riciclata la Decisione di finanza pubblica - è invece lo specchio dell'attuale impotenza politica del Governo stesso e della sua maggioranza. È, in particolare, la manifestazione della crisi politica del PDL e del suo leader, che non sono più in grado di esercitare la funzione di guida che a loro - e solo a loro - compete. Prima, nel corso dei due anni che ci stanno alle spalle, il Governo ha sostenuto, con una pervicacia degna di miglior causa, che "non si fanno riforme durante la crisi". Ora, consapevole della insostenibilità di questa linea - nel nuovo contesto europeo e globale, caratterizzato da diffuso fervore riformista - il Governo cerca in Europa, nelle scelte che saranno compiute a quel livello, quella forza politica che è necessaria per fare le riforme e che ritiene di non possedere autonomamente. Noi non possiamo costringere il Governo e la maggioranza a fare ciò che non hanno la forza di fare. Possiamo e dobbiamo però insistere sulla crescente contraddizione tra ciò che corrisponde agli interessi del Paese e ciò che il Governo - in evidente crisi politica - è in grado di offrire al Paese stesso, in termini di capacità di guida e di gestione dei problemi aperti. Sto esagerando? Governo e maggioranza hanno un modo solo per dimostrarlo: preparare una risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica che contenga prime, impegnative scelte da inserire nel Piano nazionale di riforma, la cui versione preliminare dovrà essere pronta tra pochi giorni. Noi, per parte nostra, questo faremo, a partire da questa relazione, sia pure in un contesto reso precario e difficile dai ritardi del Governo nel predisporre e presentare i documenti previsti dalla legge per la Decisione di bilancio e per le scelte di politica economica. La crisi politica in cui versano Governo e maggioranza, infatti, ha già trovato - in questi ritardi ed omissioni - significative manifestazioni. Cosa c'entra la sessione di bilancio europea con la decisione di non presentare, entro il 15 luglio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per tutto il periodo di programmazione, disfacendo così con la mano sinistra ciò che si mostra di costruire, in tema di federalismo fiscale, con la mano destra? Cosa c'entra, la sessione di bilancio europea con la mancanza, nella Decisione di finanza pubblica al nostro esame, delle indicazioni necessarie per valutare gli effetti della costruzione del bilancio a "politiche invariate" come previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *d)* - mi scuso per la pedanteria - della nuova legge di contabilità? Cosa c'entra con la sessione di bilancio europea la scelta di non indicare, come previsto esplicitamente dalla stessa legge (articolo 10, comma 2, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva? Quella indicata nella Decisione di finanza pubblica, infatti, è riportata come dato previsionale, signora relatrice, e non programmatico: un elemento di confusione che tende a caratterizzare tutte le tabelle presenti nella Decisione di finanza pubblica, malgrado la legge di contabilità sia chiarissima nel pretendere una netta distinzione tra previsione a legislazione vigente ed obiettivi programmatici. O dobbiamo intendere, signori del Governo, che, dopo la manovra di luglio, tendenziale a legislazione vigente e programmatico coincidano perfettamente? Capisco che, per tirare a campare e passare la nottata, il Governo e la maggioranza siano tentati di rispondere: sì, c'è questa coincidenza; per noi, tutto quello che c'era da decidere è già stato deciso. Ma nei panni del Governo starei attento a prendere questa scorciatoia. In primo luogo, luogo, essa confermerebbe infatti il dato di crisi politica di cui ho già parlato e l'affidamento cieco all'Europa: «tutto quel che volevamo e potevamo decidere noi l'abbiamo deciso; tutto il resto, per e su di noi, lo decideranno le istituzioni comunitarie». Per altro verso, assumendo questa posizione, il Governo sosterrebbe che programma - signor Presidente, non «prevede», sono cose diverse - il il crollo della spesa in conto capitale. Dopo la caduta del 9,7 per cento - colleghi che vi occupate di infrastrutture e che avete applaudito il Presidente del Consiglio che parlava la settimana scorsa di questo argomento in occasione del dibattito sulla fiducia

sto ripetendo le cifre di cui ha parlato la relatrice di maggioranza, forse con qualche enfasi in più col risultato di portare il rapporto tra investimenti e prodotto

le stime indicano che per ogni punto percentuale di aumento dello *stock* di capitale pubblico, cioè di investimenti in spese in conto capitale, il prodotto può crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo. E quanto alla pressione fiscale, sostenendo che il tendenziale a legislazione vigente e programmatico coincidono, il Governo mostrerebbe di programmare (e non di prevedere) un aumento un aumento della pressione fiscale fino al 2013, se si considera quella del 2009 al netto degli introiti straordinari inclusi nelle imposte in conto capitale. questo punto, il Governo non distingue tra dati tendenziali ed obiettivi programmatici semplicemente perché non si considera in grado di decidere su questi ultimi, malgrado sia perfettamente consapevole del fatto che nel nuovo contesto europeo contesto europeo non preparare con un adeguato confronto pubblico nazionale la versione preliminare del piano di riforma significa esporre il Paese al rischio di essere un soggetto passivo delle decisioni europee mentre in Europa i nostri grandi partner nell'euro fanno esattamente l'opposto. Francia e Germania (in Italia non ne sta parlando nessuno) sulla base di una decisione congiunta del presidente Sarkozy e della cancelliera Merkel del luglio scorso, stanno già procedendo - sono molto avanti - alla ricognizione dei rispettivi sistemi fiscali, con l'obiettivo esplicito di una loro rapida convergenza, con particolare riferimento - c'è scritto così nel comunicato finale - alle imposizioni sulle società, alla tassazione degli alti redditi patrimoniali, all'IVA ed alle attività elettroniche. Un primo Rapporto sulla convergenza, nell'analisi di questi due Paesi, è previsto proprio in questi giorni. Di scelte politiche di questo tipo, colleghi della maggioranza, che abbiano un carattere di vera e propria svolta, c'è oggi bisogno. È esattamente ciò che manca nella Decisione di finanza pubblica al nostro esame. Noi però e vengo alla seconda parte di questa relazione - non ci rassegniamo, così come non si rassegnano le forze sociali che rappresentano imprese e lavoratori. Mentre il Governo riduce la Decisione di finanza pubblica per il 2011-2013 a documento buono solo per i collezionisti di oggetti rari (è insieme - si legge - il primo e l'ultimo del suo genere: un oggetto da collezione) esse si riuniscono per cercare la via di una possibile fuoriuscita da una situazione di bassa crescita, di caduta della produttività, di crescente disuguaglianza, di depressione del sistema delle aspettative e di scarsa capacità di attrazione degli investimenti esteri. Per questo, malgrado tutto, ci sforziamo di entrare nel merito della Decisione di finanza pubblica, delle scelte che essa non contiene e di quelle che, a nostro giudizio, dovrebbe contenere. Partiamo dal problema della crescita troppo debole. Restiamo il secondo Paese manifatturiero dell'Unione; le nostre famiglie hanno livelli di indebitamento relativamente bassi; il sistema finanziario privato ha retto bene alla crisi; gli *stress test* hanno dato esiti confortanti. Ma abbiamo un enorme debito pubblico (ne parlerò in seguito) e da molti anni (di questo voglio parlare ora) cresciamo troppo poco: nel decennio che ha preceduto la grande recessione, la produttività di un'ora di lavoro in Italia è aumentata in media di poco più di mezzo punto percentuale l'anno, rispetto ad oltre un punto dell'area euro: sono numeri piccoli, ma 1 è il doppio di 0,5. E la produttività totale dei fattori, che stima la quota di crescita ascrivibile a fattori quali progresso tecnologico, capitale umano, miglioramento dei processi produttivi, economie di scala, cresce ancora meno: il suo livello con la crisi - è un dato impressionante - è tornato quello del 1993. Tutto ciò determina un deficit di competitività, che si traduce immediatamente in nuovi squilibri macroeconomici: da un avanzo del 3,5 del PIL nel 1996, la bilancia delle partite correnti è costantemente peggiorata e l'OCSE prevede un deficit del 3,5 per cento

Ciò che sconforta - di fronte a questi dati - è che tutti sappiamo di cosa essi sono spia, di cosa ci parlano: quindici anni di produttività stagnante sono indice inequivocabile di mercati del lavoro da riformare, fisco troppo pesante sul lavoro e sull'impresa, infrastrutture materiali e immateriali carenti, pubblica amministrazione inefficiente. Ma in tanti anni - negli ultimi dieci, ben otto governati dal centrodestra - questa comune consapevolezza non si è tradotta né in un discorso di verità al Paese, per suscitarne l'impegno e la riscossa, né in una coerente strategia di riforme strutturali: tanto "da noi si sta meglio". È anche vero. Ma chi e per quanto tempo ancora? Poiché il reddito pro-capite, al netto dell'inflazione, può crescere solo se aumenta la produttività, (questa non è una cosa né di destra né di sinistra, è un'ovvietà), la risposta che viene dai dati della realtà è la seguente: sempre meno, sempre più anziani e non per molto tempo. Anche il debito pubblico e la svalutazione della moneta sono bolle che hanno drogato il sistema: sono le nostre bolle. Ma la festa è finita. Cosa bisogna fare? La Decisione di finanza pubblica non lo dice: anzi, non si pone neppure la domanda. Ma la Strategia 2020 dell'Unione è chiara nell'individuazione dei cinque obiettivi strutturali: occupazione (la disoccupazione è finalmente considerata uno dei gravi squilibri interni della zona euro e dell'intera Unione: una vittoria postuma di quel Guido Carli che insistette invano, d'accordo con il presidente della Commissione Delors, per definire un parametro di Maastricht relativo al livello di occupazione); inclusione sociale; ricerca e innovazione; educazione; energia e cambiamento climatico. Su ognuno di questi temi, è urgente definire un'agenda delle riforme, coerente con le specificità italiane dei fattori di crisi e di debolezza, da coordinare con gli altri Paesi europei. Non si tratta di realizzare qualche aggiustamento al margine, ma di progettare cambiamenti radicali del sistema Paese. L'obiettivo è quello di un progressivo e costante innalzamento del prodotto interno lordo potenziale, cioè del livello massimo teorico di crescita che possiamo conseguire senza causare tensioni inflazionistiche. La stessa azione di rafforzamento dell'avanzo primario e di riequilibrio dei conti pubblici (ne parlerò più avanti) dovrebbe avvenire in questo contesto di riforme strutturali, in modo tale da favorire un aumento del potenziale di crescita dell'economia. Facciamo qualche esempio. L'apparato produttivo italiano, nel suo sforzo di mantenere le posizioni di eccellenza che si è storicamente guadagnato, paga un prezzo molto alto all'arretratezza del Paese nel processo di apertura del mercato dei servizi. Dall'indagine dell'OCSE in tema di regolamentazione anticoncorrenziale nei settori a rete e nei servizi professionali emerge che «i processi di liberalizzazione avviati in Italia» - sto citando alla lettera negli ultimi anni in molti comparti dei servizi si sono arrestati", per usare le parole usate da Banca d'Italia nella audizione sulla Decisione di finanza pubblica. In particolare, emerge una posizione più arretrata rispetto alla media OCSE nei comparti del trasporto aereo, della distribuzione del gas, dei servizi postali, dei trasporti ferroviari, dei servizi professionali. Mentre "è insufficiente il ruolo delle autorità di regolazione indipendenti". Queste sole valutazioni sono altrettante indicazioni di lavoro. Ma il Governo sembra muoversi Ma il Governo sembra muoversi in senso opposto: si guardi al disegno di legge sulla professione forense in discussione qui in Senato. E, soprattutto, alle strane manovre attorno ad ENI, con riferimento al gasdotto Southstream. Dall'ultimo incontro tra Berlusconi e Putin è trapelato che in quella sede sarebbero state discusse le quote di ENI e Gazprom in Southstream. Mentre lo stesso consiglio di amministrazione di ENI non ha né discusso, né deciso la partecipazione al nuovo progetto. C'è qualcosa di inquietante in questo modo di procedere. E ci sono ragioni per temere che lo squilibrio interno al mercato del gas italiano possa uscirne addirittura rafforzato. Se si guarda al mercato del lavoro, alle regole e alle procedure della contrattazione, alla qualità delle relazioni sociali, le esigenze di cambiamento sono altrettanto chiare: superare il crescente dualismo, premiare la produttività, favorire la mobilità, accrescere il livello della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, semplificare norme e procedure, anche al fine di attrarre investimenti diretti esteri in Italia. Tutto ciò, esaltando l'autonomia delle forze sociali e la loro capacità di autoregolazione, ma ma non esitando ad intervenire anche con la legge là dove il processo di modernizzazione dovesse arrestarsi in forza di insuperabili veti contrapposti. Anche a questo proposito, l'occasione della crisi rischia di andare sprecata:

Col rischio di accompagnare alla "ripresa senza occupazione" in atto in Europa l'approfondirsi del divario interno al mondo del lavoro italiano, a tutto danno, in particolare, dei giovani, delle donne e dei lavoratori impegnati nei settori esposti alla competizione internazionale.

Il cuneo fiscale sul lavoro è superiore di circa 5 punti alla media degli altri Paesi dell'area dell'euro, mentre il prelievo sui redditi da lavoro più bassi e quello sulle imprese, includendo l'IRAP, è più elevato di ben 6 punti. Un divario che deve essere superato in un contesto di pressione fiscale molto elevato in media, al limite dell'intollerabilità sui contribuenti leali, e di elevatissima evasione fiscale, particolarmente diffusa per l'IVA (circa il 30 per cento della base imponibile, oltre 30 miliardi di gettito annuo). Questo significa che la riforma fiscale deve esplicitamente essere rivolta a: ridurre le dimensioni dell'evasione fiscale, utilizzando ogni euro di gettito riveniente dal successo nella lotta all'evasione per ridurre in proporzione diretta la pressione fiscale sui contribuenti leali e in particolare sul lavoro e sull'impresa; ridistribuire il prelievo sulle diverse basi imponibili, oggi fortemente sperequato a danno del lavoro e dell'impresa e a vantaggio della rendita e della ricchezza direttamente consumata. Mi accorgo che il tempo non è sufficiente, signor Presidente, evidenziare che nella relazione scritta c'è un tentativo, cui tengo moltissimo, di collegare l'idea della lotta all'evasione fiscale, funzionale alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sulle basi imponibili del lavoro e dell'impresa, ad un'operazione di riduzione della spesa corrente primaria; senza questa seconda operazione, l'utilizzo del gettito della lotta all'evasione fiscale per ridurre la pressione sulle basi imponibili di lavoro e impresa non è credibile.

non l'ha creato la crisi, poiché le preesiste. Non è stato causa della crisi, ma costituisce un formidabile fattore di freno dello sviluppo, limita la libertà della politica economica, accentua le disuguaglianze dentro le generazioni e tra le generazioni. La sostenibilità del debito dipende dalla differenza tra crescita e tasso d'interesse. Tanto più alta è la differenza, tanto più il debito è sostenibile nel lungo periodo. In Italia, la crescita è bassa, il debito pubblico è altissimo e, per ora, i tassi d'interesse sono bassi, molto bassi. Ma per quanto tempo? Di qui l'esigenza di una svolta, che - se deve essere strutturale - deve vedere impegnato il Paese nello sforzo di ricostituire rapidamente - previo ferreo controllo dell'evoluzione della spesa corrente primaria - un significativo e permanente avanzo primario. Il ritmo della sua ricostituzione prospettato dal Governo nella Decisione di finanza pubblica è del tutto insoddisfacente: non solo per i nuovi vincoli che ci verranno posti in sede comunitaria, ma anche e soprattutto perché bisogna recuperare libertà per la politica economica e di bilancio, al fine di promuovere sviluppo e maggiore eguaglianza. In questi ultimi dieci anni l'azione del Ministro dell'economia e dei Governi Berlusconi - che oggi passano per rigoristi - ha fatto registrare il suo più grave fallimento proprio in tema di controllo della spesa corrente primaria: al ritmo di un incremento

Si può ora aggiungere un'ipotesi di lavoro che potrebbe accompagnarsi all'azione di ricostruzione di un forte avanzo primario, dandole maggiore credibilità ed efficacia: se lo Stato ha un enorme debito, ha anche un grande (quasi altrettanto grande) patrimonio. Sarebbe dunque giusto chiamare una quota di questo patrimonio - attraverso valorizzazioni e alienazioni concentrate nel tempo - a fornire un primo contributo per avviare la macchina della riduzione del debito, il cui carburante essenziale dovrebbe poi essere costituito dall'avanzo primario. È in questo contesto di credibilità e di vero rigore che non sarebbe improponibile chiedere al decile più ricco della popolazione italiana - il cui patrimonio si è molto accresciuto, nel corso di questi ultimi trenta anni, proprio mentre si costituiva l'ingente debito pubblico che soffoca il Paese - di concorrere in piccola parte allo sforzo di risanamento. il bene pubblico primario chiamato trasparenza e attendibilità dei conti pubblici. Per l'efficacia dell'azione di controllo, che ha un così grande ruolo nella nuova *governance* economica europea, «è essenziale che siano corrette che siano corrette e non politicamente inquinate le informazioni statistiche provenienti da ciascuno Stato membro, in particolare sulle finanze pubbliche». Su questo tema, saranno emesse dall'Unione europea precise raccomandazioni. Per l'Italia, si ripropone dunque l'esigenza della costruzione di una struttura tecnica di analisi economica autonoma, indipendente ed affidabile, che interloquisca con l'apparato tecnico del Governo nell'elaborazione dei dati della finanza pubblica. Ci sarà l'occasione offerta dalla immediata revisione della legge di contabilità per corrispondere all'innovazione della sessione di bilancio europea. Dobbiamo assolutamente approfittarne per reintrodurre quelle soluzioni che il Senato approvò all'unanimità durante la sua lettura della legge di contabilità, che poi la Camera cassò pressoché totalmente. Spero che quello che è accaduto nel frattempo - la clamorosa decisione assunta in proposito dal nuovo Governo del Regno Unito le raccomandazioni della Commissione - abbia convinto anche i colleghi della Camera dell'errore commesso e che ci sia oggi una nuova disponibilità a procedere, per dotare finalmente il Parlamento italiano di quell'Ufficio del bilancio unificato di cui sentiamo da tempo la mancanza, specie nella fase che stiamo vivendo di attuazione del federalismo fiscale.

nella premessa allo schema di DFP si legge testualmente che tale documento è «il primo e l'ultimo del suo genere» e che dunque, sostanzialmente, è politicamente superato. Qualche giorno fa, in occasione della riunione congiunta delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ho ascoltato con interesse alcune teorie del Ministro dell'economia, secondo le quali il fardello del debito pubblico italiano, ha raggiunto 1.843 miliardi di euro ad agosto, con una gravame di 30.716 euro per ognuno dei 60 milioni di residenti, non sarebbe un problema. Il debito pubblico è sì una pesante eredità che viene dalla finanza allegra del pentapartito ma, come si vede da uno studio elaborato da Adusbef su dati Bankitalia all'inizio e alla fine di ogni Governo, dal 1996 ad oggi cresce di più con i Governi di centrodestra. italiano era di 1170,293 miliardi di euro. Tra il 1996 ed il 2001, con il Governo di centrosinistra che ha dovuto introdurre tagli e sacrifici per raggiungere i parametri di Maastricht ed entrare nell'euro, il debito è cresciuto di 2,746 miliardi di euro al mese. Dal 2001 al 2006, dopo 58 mesi di Governo di centrodestra, il debito è aumentato di 3,824 miliardi di euro

al doppio dei Governi precedenti, con un aumento di 193,6 miliardi di euro. Queste cifre rappresentano la prova provata che i Governi di centrodestra, oltre a non avere il controllo della spesa, indebitano le nuove generazioni più degli altri. Ci sono due gravi fattori di incertezza sulla ripresa economica: l'andamento dei tassi di interesse e del costo del denaro e le politiche valutarie. Sul primo fronte, la massiccia immissione di liquidità all'interno del sistema bancario non è riuscita a rafforzarne la solidità, come dimostra il maggiore ricorso alle cartolarizzazioni da parte delle banche italiane, che oltre a non risultare più solide rispetto a quelle degli altri Paesi, dimostrano la loro rapacità a danno dei consumatori e delle famiglie. Sul ritorno dei *bankster*, che stanno trafficando sulla pelle dei consumatori e dei mercati con montagne di derivati avariati più e meglio di prima, volevo informare che non sono solo i cattivi banchieri e le banche d'affari estere ad effettuare speculazioni a largo raggio, ma anche i banchieri nostrani, che operano sulla pelle delle famiglie, come dimostra un recente studio del commissario europeo ai servizi finanziari Michel Barnier.

considerare una serie di aumenti. Non si capisce perché il Governo non intervenga per calmierare la rapacità dei banchieri, che continuano a vessare e strangolare le famiglie, le piccole e medie imprese, con una forbice di 14 punti sui tassi, pari allo 0,04 per cento sui depositi e al 14,5 per cento sugli impieghi, con richieste di 5,8 euro per pagare una bolletta allo sportello o di 8,5 euro per un bonifico. L'andamento della finanza pubblica imporrebbe un'immediata analisi dei principali capitoli di politica economica, come l'aumento della disoccupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie e degli investimenti nel settore edilizio, una consistente diminuzione dei contributi sociali e dei redditi da lavoro dipendente DFP come principali fattori della generale flessione delle entrate - il mancato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che avrà un impatto economico negativo sul mondo del lavoro. Lo schema di DFP risulta insoddisfacente sul fronte tributario, non recando al suo interno alcun riferimento alla riforma del fisco e all'introduzione del quoziente familiare. La crisi, signor Presidente, non è stata ancora superata, come si evince dal più recente rapporto OCSE, pubblicato ieri, sull'andamento della congiuntura nei 30 Paesi membri, che ad agosto evidenzia il rafforzamento dei segnali di rallentamento della crescita già apparsi negli ultimi tre mesi, particolarmente forti per Canada, Francia, Italia, Regno Unito, Brasile, Cina e India e ancora peggiori per gli Stati Uniti (Germania, Giappone e Russia sembrano invece continuare nella fase espansiva). ad agosto 2010 erano senza lavoro 45,5 milioni di persone, 13,4 milioni in più rispetto al luglio 2008, a conferma che da questa crisi prodotta dai banchieri e dagli omessi controlli delle autorità vigilanti colluse, che regalano denaro alle banche fornendo loro formidabili munizioni per speculare, a perderci sono stati i lavoratori, le famiglie e la maggioranza delle popolazioni. Certo, ci sono poi anche quelli che hanno guadagnato dalla crisi. I patrimoni detenuti dai privati nel mondo sono saliti del 72 per cento negli ultimi dieci anni nonostante la devastante crisi economica scoppiata nel 2007, ma le disuguaglianze, seppure in diminuzione grazie alla crescita di Cina e India, restano abissali. Appena l'1 per cento della popolazione mondiale possiede il 43 per cento delle ricchezze private e, alla base della piramide, il 50 per cento delle persone solo il 2 La gran parte della ricchezza è concentrata in Europa e in Nord-America. Nonostante un decennio di rendimenti reali vicini allo zero sui titoli azionari e lo scoppio delle bolle immobiliari, i patrimoni posseduti dai privati nel mondo sono, ripeto, saliti del 72 per cento restano le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, tuttavia l'India, in fondo alla classifica, ha raddoppiato il dato del PIL per abitante negli ultimi dieci anni, mentre Cina, Romania e Polonia hanno visto triplicare i propri risultati. Ci sono eccezioni come Islanda ed Argentina, finite in bancarotta (meno 30 per cento), o come Giappone e Stati Uniti, dove la crescita è stata esigua. Nel dettaglio, la ricchezza detenuta dagli individui è cresciuta dalla media di 30.700 dollari nel 2000 43.800 dollari nel 2010, con un aumento del 43 per cento, che sale al 72 per cento considerando l'incremento della popolazione globale mondiale da 3,6 a 4,4 miliardi di abitanti. Una media che mette posizioni distanti, come i 250.000 dollari di Svizzera, Norvegia o Francia, insieme a quelle di Paesi con meno di 5.000 dollari, quali India, Bangladesh e quasi tutti gli Stati dell'Africa centrale o occidentale. Circa 3 miliardi di persone nel mondo (due terzi del totale) hanno una ricchezza sotto i 10.000 dollari, mentre alla sommità della piramide circa 81.000 persone nel mondo hanno un patrimonio sopra i 50 milioni di dollari. L'Italia, signor Presidente, si piazza ai primi posti della classifica mondiale, con un raddoppio dei patrimoni nel decennio, anche se gran parte della ricchezza (il 60 per cento) è costituita dal patrimonio immobiliare, e il debito medio è di 21.000 dollari, appena il 9 per cento dei

I "Paperoni", ovvero coloro che possiedono un patrimonio sopra un milione di dollari, in Italia sono 1,4 milioni, e così 2,8 milioni di italiani appartengono a quella fascia dell'uno per cento di fortunati nella piramide della ricchezza mondiale. Ho citato questi dati, signor Presidente, perché questo è un Governo che non ha fatto nulla negli ultimi anni per fare in modo che queste disuguaglianze sociali e questi gravissimi squilibri venissero in un certo modo azzerati, ma anche perché di fronte a questi dati diventa ancora più urgente l'armonizzazione delle aliquote fiscali (non abbiamo visto nulla di questo) sulle rendite finanziarie che, salvaguardando tutti i titoli di Stato, possa finalmente far pagare quei "Paperoni" e quegli speculatori che versano la stessa ritenuta alla fonte, ossia il 12,5 per cento, come gli operai ed i comuni cittadini che fanno fatica per mettere da parte i sudati risparmi investiti in BOT e BTP. Per queste ragioni, signor Presidente, diamo un giudizio molto negativo su un Governo che fa finta di litigare con i banchieri ma poi ci va a braccetto;

concentrerò il mio intervento esclusivamente sul documento Allegato infrastrutture, essendo questo tradizionalmente il principale atto di programmazione riguardante gli investimenti in infrastrutture; un atto sul quale la Commissione competente di questa Camera si esercita come di consueto nelle proprie considerazioni. In questo ultimo decennio molte sono state le novità sul piano amministrativo, contabile e politico per fare di questo appuntamento un'occasione di innovazione di questo essenziale strumento: dall'alternanza delle maggioranze politiche e di Governo che si sono succedute, alle riforme contabili, ai mutati assetti che i Dicasteri hanno conosciuto. Di volta in volta in volta si è cercato di conferire un taglio, almeno nella parte analitica del documento, che potesse essere in grado di conferire un'impronta significativa e duratura ad un tema tanto complesso e vischioso come quello legato alla programmazione degli investimenti. Si è trattato di tentativi - possiamo dirlo con buona pace per tutti - miseramente falliti alla prova dei fatti. Su questo altare è stata immolata perfino la cosiddetta Legge obiettivo, che nelle vostre intenzioni, colleghi della maggioranza, avrebbe dovuto essere risolutiva nella concentrazione delle risorse e nell'accelerazione delle procedure e dei tempi di realizzazione. Purtroppo, è stato tristemente vero il contrario: i tempi di realizzazione si sono dilatati e le risorse si sono disperse; ma mai avremo immaginato di assistere a un tentativo, come quello oggi in esame, di fatto abortito ancor prima di nascere. Si tratta di un documento che ha visto l'assoluto disinteresse nello stesso Governo e dello stesso Governo, che non è venuto neppure a presentarlo in Commissione e che ha visto registrare la distanza da parte della stessa maggioranza parlamentare. Faccio notare, signor Presidente, che la Commissione di merito non ha neppure espresso il parere relativo, non ho ancora capito se per carità di Patria o per reale disinteresse. L'Allegato infrastrutture infatti, al di là delle tabelle su cui di anno in anno si registrano gli scostamenti tra le intenzioni dichiarate e le risorse reali effettivamente disponibili, costituisce un momento per rappresentare anche materialmente l'idea di sviluppo per il Paese che si intende perseguire con l'azione di Governo. È l'occasione principe per consegnare al Parlamento e al Paese la visione che si vuole offrire e la missione che si intende perseguire nell'ammodernamento infrastrutturale per rafforzare l'economia del sistema Paese. Purtroppo dispiace constatare che il documento nient'altro è che un *patchwork*, un lavoro fatto di pezzi assemblati, privi di un collegamento organico, occasione tutt'al più per qualche invenzione retorica pensata appositamente per gli effetti mediatici, ormai privi di credibilità sull'argomento. Anche le migliori intenzioni rappresentate sortiscono l'effetto di un trucco che non funziona più, tanta è la distanza tra i concetti espressi e la cruda realtà che anche i cittadini ormai percepiscono. La stessa composizione disorganica del documento tradisce le reali volontà di un Governo e di una maggioranza, che evidentemente preferiscono derubricare questo dibattito a mera e stanca ritualità parlamentare, a cui loro malgrado non si possono negare. Per questo la sensazione più forte che avvertiamo è che in fondo ci troviamo nel paradosso di prendere sul serio un documento che voi stessi avete prima ritardato e poi evitato di esporre ad un confronto di merito nella Commissione competente. Il motivo è al contempo molto semplice e abbastanza grave: al di là delle buone intenzioni, che non mancano mai in ogni documento e in ogni proposito, questo fondamentale atto di programmazione manca degli essenziali requisiti. Manca un'effettiva trasparenza nell'indicazione delle risorse e una reale selezione delle priorità negli interventi che si intende veramente perseguire. Non sono innanzitutto chiare nel documento le risorse effettive oggi disponibili e si ricorre infatti, non a caso, ad un forma retorica quanto meno singolare, parlando in proposito di risorse «potenzialmente disponibili»: si tratta di un lessico che già la dice lunga sulla reale disponibilità delle risorse indicate. modo non sono chiare le risorse disponibili in prospettiva, specie quelle per le quali si segnala da tempo l'impiego di risorse private, ma che puntualmente registrano opere di fatto rimaste al palo. Non sono chiare neppure le risorse che sono state impiegate in questi anni e il reale stato di avanzamento delle opere. Si citano percentuali realizzative a casaccio, o si fanno affermazioni generiche di dubbia attendibilità. La prova più eloquente l'abbiamo avuta ed è stata probabilmente quella che ci hanno offerto il Presidente del Consiglio prima - proprio in quest'Aula - e il Ministro delle Infrastrutture poi con una nota a parziale rettifica, nelle loro convulse e affrettate dichiarazioni a proposito dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Molto probabilmente e più semplicemente non si sono presi neppure la briga di leggere o di farsi riferire che cosa veniva scritto dai loro stessi funzionari Per il 2013, infatti (è bene ripeterlo in anticipo e a chiare lettere) la Salerno-Reggi Calabria non solo non sarà completata per il 90 per cento, ma se le cose andranno proprio bene non sarà conclusa neppure per il 60 Suggerisco al Ministro di farsi aggiornare con i cronoprogrammi ANAS sull'effettivo stato di avanzamento dei lavori e non di quelli appositamente fermati da due anni a questa parte. Sappiamo bene che la situazione finanziaria del nostro Paese è appesantita in maniera insopportabile da un debito pubblico, che tutti abbiamo prodotto e per il quale dobbiamo chiedere tutti scusa alle nuove generazioni. Un debito che tarpa le ali oltre che a loro, anche ad ambiziosi ma necessari programmi di investimento per la realizzazione di opere strategiche fondamentali per il Paese. Ma proprio per questo l'imperativo categorico per chi è chiamato dalla volontà popolare ad amministrare le risorse pubbliche nell'interesse della collettività, dovrebbe essere quello di avere a cuore un'attitudine a selezionare le priorità strategiche per concentrare su quelle le risorse effettivamente disponibili. Si assiste, invece, drammaticamente all'opposto, con l'indicazione di opere di dubbia rilevanza strategica (una su tutte il Ponte sullo Stretto) o all'elencazione di opere i cui costi e i relativi tempi di realizzazione sono allo stato dell'arte assolutamente improbabili. È così per la Napoli-Bari (nessuna risorsa, costo stimato almeno 5 miliardi di euro); ed è così per la Ionica

alpini e, ancora, dell'Expo 2015, la cui realizzazione delle opere è soltanto circoscritta agli interventi finanziati dal Governo precedente, mentre per quelle che dovevano essere aggiunte sicuramente non ci sarà nessuna realizzazione per l'inizio dell'evento. Ma allora cosa aspettiamo a riformare davvero in maniera trasparente questo Paese, che voi state bloccando in un incomprensibile immobilismo politico, proprio quando sarebbe necessario un colpo d'ala per evitare il precipizio a cui un lento ma inesorabile declino lo sta conducendo? Già prima di me nella relazione di minoranza sono state indicate le priorità che potevano e dovevano essere colte con questo provvedimento. A partire dal recupero di produttività del sistema Paese, ad un credibile abbattimento del debito pubblico, ad un processo di riforma che guarda all'apertura vera dei mercati e al fattore della concorrenza regolata come unico strumento in grado di scardinare anacronistiche posizioni di rendita monopolistica, presenti in tutti i principali settori economici del Paese. Una situazione, quella dell'Italia di oggi, che di fatto ostacola anche la possibilità di determinare l'attrazione di capitali privati e stranieri. Nel documento queste cose sono indicate tra le righe, verrebbe da dire di mala voglia. Viene da dubitare che siano state scritte senza neppure la reale consapevolezza del Ministro. Se così non fosse, chiedo scusa, ma lo invito a procedere con coerenza e trasparenza in questi propositi, a fare presto e bene perché il Paese non ha più tempo da perdere, ne ha perso fin troppo in tutti questi anni. Saremo vigili e scrupolosi osservatori, a partire dalla liberalizzazione del sistema ferroviario: disponga il Ministro gli atti necessari per procedere; a partire da un'effettiva autorità indipendente, come gli è stato anche recentemente chiesto, utilizzando magari anche una tra quelle esistenti: proceda allo scorporo societario della rete ferroviaria dalle società di gestione dei servizi. Infine, estenda il processo di liberalizzazione anche al servizio universale, magari - ci permettiamo di suggergli - creando un'apposita società per l'affitto del materiale rotabile. Dia davvero seguito alla volontà del Parlamento, recentemente manifestata anche in questa Aula e presente nella legge di riforma, di disporre per i porti, che rappresentano strutture davvero strategiche per il rilancio dei traffici nel Paese, l'autonomia finanziaria degli scali finalizzata alla realizzazione di quelle infrastrutture indispensabili al loro rilancio, a partire dai dragaggi per l'approfondimento dei fondali e dai collegamenti ferroviari all'Alta Velocità, trasformandola compiutamente - come voleva il progetto originario - in Alta Capacità. Venga intanto però il Ministro delle infrastrutture in Commissione a riferire su come, nel frattempo, avrebbe dovuto riadeguare la politica degli investimenti a seguito del taglio di 3 miliardi e 300 milioni intervenuto con la finanziaria 2010; tagli operati dal suo collega ministro Tremonti, non dal precedente Governo. È da gennaio che ne reiteriamo costantemente la richiesta; lo stiamo ancora aspettando. Ci raccomandiamo al riguardo anche alla Presidenza, affinché se ne faccia autorevole interprete. E soprattutto il Ministro faccia tirare fuori dal cassetto in cui è riposto il piano degli aeroporti (che in questo documento è soltanto appena accennato) e lo venga a presentare, quando vuole, peraltro dovuto, alle Commissioni parlamentari di merito. Su quello, non su nessuna copia artefatta, potremmo anche essere disponibili all'adeguamento delle tariffe aeroportuali, ferme da tempo, per finalizzarle alle sole infrastrutture prioritarie che in quel documento sono indicate. Purtroppo, abbiamo il timore che così non sarà, perché così non volete che sia.

parlo di disarmante onestà. Già nelle prime cinque righe di quel documento c'è scritto che, sostanzialmente, il titolo non corrisponde ai contenuti, in quanto non contiene nessuna decisione di finanza pubblica; onestamente che questo è, o avrebbe dovuto essere, il primo documento di Decisione di finanza pubblica rispetto alla riforma che abbiamo varato per la legge di bilancio, ma, così com'è quest'anno, è anche l'ultimo, perché i prossimi documenti dovranno essere scritti di concerto con l'Europa. Perché è di una disarmante onestà? Perché sostanzialmente si scrive, in termini di decisioni di finanza pubblica, che le decisioni che avrebbero dovuto essere prese nella sessione di bilancio di quest'anno sono già state prese e anticipate con la manovra di luglio. Peraltro, le decisioni che dovranno essere prese in prospettiva dovranno essere prese nel futuro in coerenza con il nuovo quadro europeo delle decisioni strutturali definite in sede europea. Anche il collega Morando ha fatto notare che una prima scadenza, da questo punto di vista, è proprio nel mese di novembre, quando l'Italia, come gli altri Paesi, dovrà presentare in sede europea quelle linee di politica economica. Vorrei approfondire il mio ragionamento per cui il documento, di fatto, non contiene decisioni di finanza pubblica, tanto da riprodurre esattamente, negli stessi numeri, tutte le tabelle che sono state già pubblicate

essendo stata anticipata, rende inutile la legge finanziaria per il 2011, tanto che quest'ultima legge viene anticipata come una legge puramente tabellare. Come ha ricordato la relatrice Bonfrisco nella sua relazione (e questo lo si può leggere - per questo è di una disarmante onestà,

ciò che tutti noi abbiamo deciso con quella manovra di luglio (e che personalmente condivido profondamente), si pone da una parte l'obiettivo di tagliare

Quindi, sottoscrivendo pienamente quell'obiettivo, avevo già avuto modo e occasione di dire che purtroppo, però, il perseguimento dello stesso è realizzato con una strategia di politica economica che riguarda i livelli e la composizione, sia della spesa sia delle entrate - e non il puro saldo finanziario - che in realtà generano effetti controproducenti, nel senso che frenano la crescita e dunque indirettamente, in prospettiva, rendono più precario l'obiettivo stesso del raggiungimento del riequilibrio del deficit pubblico. In occasione di quella manovra, il Servizio studi del Senato nel

oltre al taglio del deficit, abbiamo deciso di aumentare la spesa corrente di 26 miliardi, di ridurre gli investimenti di 3 miliardi e di aumentare le entrate di 48 miliardi: se si confrontano i dati con quelli veri, rispetto al dato storico di quest'anno, perché il taglio sui tendenziali è riferito a numeri nei prossimi anni che non esistono ancora nella realtà economica. Dunque, dopo quei tagli tendenziali, se si confrontano quei tagli con il dato storico di oggi, questo è il risultato: abbiamo aumentato la spesa corrente di 26 miliardi, ridotto il valore assoluto degli investimenti di 3 miliardi e aumentato le entrate di 48 miliardi,

e, come la relatrice Bonfrisco ha chiaramente indicato, questa tendenza prosegue anche negli anni futuri, in cui non viene contenuta

in collegamento con l'Europa per il 2015 e il 2016. Ma l'Europa giustamente guarda i saldi finanziari e lo *stock* di debito pubblico,

qualche Paese europeo potrebbe essere interessato ad un'Italia che si indebolisce strutturalmente, continuando però a garantire i saldi finanziari, perché sul piano della competizione reale, della produzione, forse un'Italia più solida e più forte può anche dar fastidio.

Anche il nostro Gruppo ha, ovviamente, dato la fiducia al Presidente del Consiglio proprio su quei cinque punti, che sono cinque punti del programma elettorale sul quale si è manifestato il

sicuramente non nella prossima legge finanziaria, ma nulla in attesa del quadro europeo. Signor Presidente, Signor Presidente, spesso, negli anni passati, da molte parti si è usata la difficoltà della situazione economica internazionale e della crisi finanziaria. Ricordo che nel 2001 vi fu il crollo delle Torri questa volta c'è la crisi economico-finanziaria internazionale. Bene, qualcuno interpreta la situazione di crisi esterna all'Italia come la impossibilità, data la crisi, di procedere alle riforme strutturali che la maggioranza si è impegnata a realizzare di fronte agli elettori. Io sono di opinione totalmente opposta. Quelle riforme strutturali l'Italia le avrebbe dovute fare da anni, ma proprio perché c'è la crisi economica internazionale, proprio perché ci sono fibrillazioni sui mercati finanziari, a maggior ragione è urgente che il Paese, nella sua parziale e ridotta autonomia decisionale di politica economica, adotti quelle riforme profonde di cui ha bisogno per affiancare la gamba del rigore finanziario. Tale gamba, ineludibile (e chiunque affermi il contrario sarebbe un irresponsabile in termini di un solo euro in più di *deficit* pubblico o di debito), è una gamba insufficiente se non si affianca a quella delle riforme strutturali a sostegno della crescita e dello sviluppo. Signor Presidente, io ho avuto l'onore di avere grandi maestri economisti.

il mio maestro Robert Solow, premio Nobel, ha prodotto una teoria economica consolidata da 40 anni, non discussa da nessuno nell'ambito degli economisti. Questa teoria sostiene che, se il tasso di interesse è maggiore del tasso di crescita economica, il rapporto tra debito e PIL è destinato ad esplodere. E i mercati finanziari che anticipano queste cose, queste cose le sanno. Se il tasso di crescita è superiore al tasso di interesse, Se il tasso di crescita è superiore al tasso di interesse, il rapporto tra debito e PIL è invece destinato a ridursi.

in questo momento siamo fortunati, perché i tassi reali di interesse sono quasi pari a zero e, da questo punto di vista, siamo in una congiuntura particolarmente favorevole. Ma sappiamo tutti che che i tassi di interesse sono destinati ad aumentare nei prossimi anni e, non appena il tasso di interesse supererà quello striminzito, asfittico tasso di crescita, i mercati percepiranno immediatamente che

crescita mondiale, crescita italiana, tassi di interesse, tassi di cambio. Lì, in quelle tabelle, c'è un euro a 1,30 e a 1,35, ma Dio non voglia che l'euro vada a 1,45, perché si dimezzerebbe il tasso di crescita dell'economia italiana.

grande crisi internazionale. Se non ci sarà rapidamente una nuova *governance* mondiale - timidamente apparsa a Washington con la mia vecchia idea di cinque anni fa di chiedere alla Cina la flessibilità del renminbi cinese

di essere stati la ricarica di una grande molla di crisi. Abbiamo una finestra di opportunità, come Italia e come Europa. Questo è il momento di sfruttare tale finestra di opportunità; non è il momento di rinviare ulteriormente decisioni,

la nuova legge di contabilità impone all'Esecutivo, come è noto, l'obbligo di presentare lo schema di Decisione di finanza pubblica entro il 15 settembre di ogni anno, al fine di consentire alle Camere di esaminare in tempi congrui i contenuti e stabilire l'entità della successiva manovra finanziaria nonché le cifre e le modalità attraverso cui questa entità si raffigura nei saldi di finanza pubblica. Lo schema di Decisione di finanza pubblica è stato invece presentato alla Camere ben oltre il termine stabilito dalla legge di contabilità pubblica, violando così una prerogativa del Parlamento e precludendo allo stesso la possibilità di un approfondito esame del quadro programmatico e dell'efficacia degli obiettivi, peraltro non chiaramente rinvenibili. L'irrilevanza politica poi del documento deriva da un'ulteriore duplice circostanza. Da un lato, la manovra di finanza pubblica è stata anticipata a luglio e, giacché l'Esecutivo persevera nell'atteggiamento di scegliere di non scegliere, l'effetto del decreto legge n. 78 del 2010 sulla crescita del PIL deve ritenersi di segno ampiamente negativo, con conseguenze che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita dì competitività complessiva del Paese. Inoltre, l'ormai imminente approvazione del nuovo Patto di stabilità e di crescita a livello europeo impone di procedere ad una disamina politica, anziché meramente tecnica, del contenuto della Decisione di finanza pubblica. Infatti, il 29 settembre, lo stesso giorno in cui il Presidente del Consiglio si presentava alla Camera per chiedere il voto di fiducia, la Commissione europea approvava il pacchetto di misure sulla *governance* economica. L'obiettivo è una migliore sorveglianza delle politiche di bilancio, delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali degli Stati membri, attraverso nuovi meccanismi di controllo quali, in particolare: il rafforzamento del Patto di stabilità e di crescita; la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; la cronologia e una panoramica del nuovo sistema di sorveglianza ed implementazione. A fronte dei suddetti elementi, la proposta della Commissione europea prevede inoltre che il nostro Paese debba, nei prossimi 10 anni, procedere ad una drastica, consistente, massiccia, rilevantissima riduzione del debito pubblico con aggiustamenti che prevedono manovre economiche di portata obiettivamente epocale. Tutto ciò per tentare di riportare il nostro debito pubblico al 60 per Con gli attuali tassi di interesse e gli scenari di crescita della nostra economia, che vengono da tutti condivisi, questo aggiustamento comporterà prevedibilmente un avanzo primario di circa il 5 per cento del prodotto interno lordo. Questo è un obiettivo impegnativo, e la Decisione di finanza pubblica contempla però avanzi primari mediamente inferiori al 2 per cento per i prossimi tre anni e si limita a stabilizzare il debito ai livelli del 2009, non certo a ridurlo. Quindi, si prospetta una manovra complessivamente di circa 9 punti di PIL in 3 anni. Se questa riduzione del debito non verrà conseguita da qui a tre anni il nostro Paese dovrà pagare una sanzione che potrebbe ammontare a più di un punto di PIL cento più un decimo dello scostamento, quindi lo 0,9 per cento per un totale dell'1,1 per cento del prodotto interno lordo). Il Governo, se intende rispettare questi impegni, deve quindi modificare profondamente l'indirizzo di politica economica sin qui seguito, puntando su una più forte crescita della nostra economia e su interventi di contenimento della spesa pubblica e di contrasto all'evasione fiscale ben più incisivi di quelli varati sinora. Eppure nella Decisione di finanza pubblica non vi è cenno ad una strategia di rientro del debito pubblico. Negli interventi alla Camera e al Senato del Presidente del Consiglio, alla richiesta del voto di fiducia, nessuna parola è stata spesa su tale argomento. Non si è ritenuto, insomma, di comunicare direttamente agli italiani questi impegni gravosi che si stavano prendendo a livello europeo. I casi sono tre: o il Governo è convinto di non farcela a sopravvivere da qui alla fine della legislatura, e dunque è intenzionato a scaricare la "patata bollente" al prossimo Esecutivo, Esecutivo, o conta su una non applicazione di queste regole, oppure conta di ridurre solo il debito lordo, ma non il debito netto. Appare quindi oltremodo pericoloso proseguire lungo la strada dello svuotamento del dibattito sulla politica economica e di finanza pubblica: l'entrata in vigore nel 2016 del nuovo Patto europeo di stabilità e crescita imporrà anche al nostro Paese un percorso di rientro dal proprio debito particolarmente gravoso, nel presupposto di una crescita economica particolarmente modesta. Sono pertanto ingiustificate da questo punto di vista le accuse di catastrofismo rivolte a quanti sollevano tali questioni. Il Governo ha al contrario il compito di delineare immediatamente una strategia di riallineamento della propria programmazione economico-finanziaria per non farsi trovare impreparato rispetto all'introduzione dei nuovi vincoli europei, per dovere di onestà politica ed intellettuale. l'andamento della finanza pubblica impone un'analisi immediata dei principali capitoli di politica economica, come l'aumento della disoccupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie, il permanere inoltre di un grave squilibrio dei conti pubblici, a testimonianza del fallimento delle politiche economiche del Governo. I dati relativi all'andamento della finanza pubblica per il 2010 confermano peraltro le gravi difficoltà esistenti. Spiccano, al riguardo, i preoccupanti dati programmatici relativi all'andamento del debito pubblico previsto nel 2010 al 118,5

l'inefficacia delle misure di stabilizzazione automatica delle spese e l'assenza di credibili riforme strutturali per il Governo della spesa. Inoltre, l'avanzo primario, principale indicatore del buon andamento della finanza pubblica, è stato completamente eroso nel corso degli ultimi due anni, registrando un disavanzo dello 0,3 per cento nell'anno in corso. Nel documento al nostro esame, l'Esecutivo prefigura un percorso di risanamento finanziario che produrrà una correzione dell'andamento con un avanzo per il 2011 dello 0,8 Ad aggravare il quadro di finanza pubblica, la DFP stima per il 2010 un forte calo del gettito delle entrate tributarie da imposte dirette, pari a circa 7,156 miliardi di euro rispetto alle previsioni della RUEF 2010, e per 8,186 miliardi di euro nel 2011. Le entrate totali, come riferisce la DFP, registrano un contenimento della loro incidenza rispetto al PIL che passa dal 47,2 per cento nel 2009 al 46,4 per cento A fronte del forte calo delle entrate tributarie da imposte dirette, la DFP registra comunque un andamento della pressione fiscale che raggiunge nel 2010 il 42,8 per cento in rapporto al PIL, rimanendo per tutto il periodo del quadro programmatico di previsione significativamente al di sopra del 42,4 Le stime della DFP sulla crescita economica, poi, evidenziano per l'anno 2010 una crescita del PIL dell'1,2 per cento, superiore alle più recenti stime dell'OCSE e dell'UE, ed una crescita dell'1,3 per cento nel 2011, ben al di sotto delle previsioni di crescita del resto dei Paesi dell'Unione e di quelli maggiormente sviluppati. Una crescita così bassa è fonte di forte scetticismo circa l'efficienza delle politiche programmatiche per lo sviluppo e tale da far sembrare irrealizzabili gli obiettivi di finanza pubblica. In sintesi, la DFP, visti i dati sull'andamento economico e finanziario, presenta un quadro da cui emerge chiaramente una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto in base all'andamento del ciclo economico ma, al contrario, come un deterioramento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro. Difficoltà che ci impediscono di agganciare il treno della ripresa, così come stanno facendo il resto dei Paesi maggiormente sviluppati, e ci condannano ad andare a loro rimorchio. La gravità della situazione in cui si trova l'Italia non può più essere attribuita per intero e soltanto agli effetti della crisi economica e finanziaria internazionale. Al contrario, in proposito, molto dipende, ed è dipeso, dall'immobilismo del Governo e dalla reiterata sottovalutazione dei problemi del Paese.

Ci chiediamo al riguardo dove sia finita la riforma del sistema fiscale, dove sia finita l'introduzione del quoziente familiare. Nulla di tutto ciò è menzionato nello schema di Decisione di finanza pubblica. Eppure queste priorità sono state indicate come punti qualificanti del programma politico sul quale il Governo ha recentemente ottenuto la fiducia delle Camere. Anche questo fa parte del fallimento della politica degli annunci, come il proclamato Piano per il Sud. Solo un dato per tracciare un quadro, purtroppo definitivo, sul tema. Nonostante la flessione, in valori assoluti il PIL ai prezzi di mercato per abitante del Centro-Nord continua ad essere sensibilmente più elevato di quello del Mezzogiorno: 30.036 euro nel Nord-Ovest, 29.746 euro nel Nord-Est e 28.204 euro nel Centro, contro i 17.324 euro del Mezzogiorno. In questo contesto, non una parola, né nella Decisione di finanza pubblica, né in quant'altro che ci faccia capire come si esce da questa spirale e da questo circolo assolutamente poco virtuoso.

la panacea di tutti i mali e che avesse risolto i problemi della legge finanziaria. Ricordate il dibattito sulla legge finanziaria? Ci siamo ridotti alla circostanza che facciamo una finanziaria ogni tre mesi, senza avere un quadro d'assieme delle politiche economiche e finanziarie del Paese. Credo che questo documento, che dal nostro punto di vista ha un valore, certifichi il fallimento della politica economica e finanziaria del Governo, che deve radicalmente cambiare rotta.

Per rubare l'affermazione di un collega che ha parlato poco fa, non so se siamo di fronte ad una disarmante onestà o, al contrario, ad una pericolosa, pericolosissima incapacità,

sta approssimando un nuovo appuntamento, che è ormai vicinissimo (il senatore Morando ricordava una scadenza del prossimo mese di novembre), nel corso del quale, nell'ambito del nuovo Patto di stabilità e di crescita, l'Europa verrà in nostro per farci decidere ciò che non riusciamo a decidere. Attenzione, però: quando si decide in questo modo decidono gli altri per noi. E se decidono gli altri per noi, non è affatto detto che le decisioni che verranno assunte vadano nella direzione degli interessi che comunque nell'ambito dell'Unione europea noi dobbiamo sempre tutelare, cioè gli interessi del nostro Paese, dei cittadini italiani, che essendo appunto cittadini di un Paese fondatore non possono sostenere una situazione e un quadro di questo tipo. Il quadro internazionale, come è stato ricordato, mette in evidenza due aspetti fondamentali, almeno dal mio punto di vista. Il primo è che l'Italia, con la sua debole crescita, tiene giù l'Europa e che l'Europa, ahimè, con la sua debole crescita tiene giù il mondo.

elevate di quelle che si registrano nel complesso dell'Europa. Questi sono due elementi di riferimento di quadro e di contesto internazionale con i quali non si può fare a meno di misurarsi per cercare di individuare quali soluzioni in Europa e, dentro l'Europa, in Italia, possiamo provare a mettere in campo per evitare di continuare ad essere il fanalino di coda di una crescita mondiale alimentata, come sappiamo, prevalentemente dall'Asia e dall'America meridionale. Ora, in questo nuovo quadro di governo europeo della finanza pubblica, il problema principale che dovremo affrontare - penso preventivamente e non a consuntivo, come invece pare voglia fare il ministro Tremonti

verso la crescita, e soprattutto garantire la stabilità. Tutta qui sta la differenza, e attorno a questo tema si confronteranno i Paesi dell'Unione, con le loro diversità, per vedere se riescono a determinare una *governance* politica comune

non che le altre siano meno importanti - è come sia possibile, come dicevo prima, correggere tutti questi elementi di debolezza, che sono prima italiani e poi europei, perché il vecchio continente

credo noi in Europa dobbiamo discutere davanti ai problemi che la situazione internazionale ci propone. In questa situazione il problema è il debito, come abbiamo detto, e la produttività del sistema, inteso nella sua dimensione più larga. Ci siamo dati degli obiettivi, come la riduzione del disavanzo al 2,2 per cento nel 2013, individuando soltanto due terreni di azione: il taglio delle spese, come abbiamo già fatto con la manovra di luglio, e la lotta all'evasione. Io considero questi due strumenti individuati assolutamente insufficienti per raggiungere tale obiettivo, così come vengono dichiarati. Penso che la lotta all'evasione non possa essere separata da un ripensamento complessivo del sistema di prelievo fiscale e soprattutto da una condivisione con gli altri Paesi dell'Unione del sistema di prelievo fiscale. In sostanza, gli obiettivi che questo documento ci propone sono una grande fatica per tornare ai livelli del debito del 1998: cioè, nel 2012 raggiungeremo una quota del 115,2 per cento che, ahimè, era esattamente la situazione che si era determinata nel 1998, sapendo che la riduzione che ci verrà proposta dal nuovo Patto di stabilità, se non cambiano le regole, come dice la formuletta sulla quale si è già raggiunta un'intesa, ci imporrà il 2,9 per cento all'anno di riduzione rispetto al PIL del debito che abbiamo. Questa, come sappiamo, è una cifra che ha una dimensione rilevantissima, a consuntivo e non invece valutando le misure da adottare in maniera preventiva. Abbiamo esplorato molte strade per cercare di ridurre il debito: abbiamo immaginato di mettere a valore il patrimonio, come pure una modifica del sistema fiscale che fosse contemporaneamente capace di ridurre l'evasione e di introdurre delle novità. Non credo

Non esistono soltanto i fondi sovrani, ma anche la speculazione sovrana che ovviamente si può permettere chi ha concentrato in un solo punto tutte le manovre di politica

quale sono attualmenteabituati. Siamo alle prese con decisioni di una portata tale che richiederebbero una maggioranza politica solida e, in quanto tale, capace di convenire con l'opposizione una "linea Paese"

presentati, siamo molti lontani da questa situazione e non vedo all'orizzonte un tempo che ce la faccia raggiungere come sarebbe necessario.

Piace anche a me ricordare i cinque grandi obiettivi della Strategia europea 2020, che sono l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, l'energia e la povertà: cinque grandi temi che ci dovranno vedere impegnati a pieno titolo e a pari livello con gli altri *partner* europei. Vi sono alcuni documenti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Europa e nostra. Per quanto riguarda lo *Stability Programme*,

Per quanto concerne il *National Reform Programme*, sussistono problematiche da affrontare, poiché l'Italia ha un debito pubblico molto elevato (il terzo in Europa) e deve impostare e far approvare dall'Unione europea un programma proiettato nel decennio 2010-2020 che contenga interventi di politica economica idonei a ridurre il debito pubblico e, nel contempo, a creare i presupposti di crescita e competitività economica in linea con la politica europea.

un piano di grandi infrastrutture che sia coerente ed interconnesso, considerato che spesso si sviluppano dei particolarismi che non sono efficienti ed efficaci per gli interessi generali.

concreta e vera ai bisogni delle famiglie e delle imprese. La DFP si propone, pertanto, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, di mantenere il controllo sul disavanzo pubblico attraverso una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella corrente primaria. Ricordo che la spesa pubblica, al netto degli interessi, sarà ridotta di 4 punti percentuali passando dal 47,8 per cento del 2009 al 43,8 per cento

Il processo federale garantirà la stabilità finanziaria in coerenza con i nuovi meccanismi dell'area euro e le nuove regole del patto rafforzato di stabilità e crescita europeo. Sarà l'unico strumento legislativo idoneo a superare le anomalie di funzionamento e le inefficienze di spesa prodotte dall'attuale sistema di fiscalità delle autonomie territoriali. completare l'attuazione del federalismo fiscale, come chiave per ristabilire e rilanciare il patto su cui si fonda l'unità nazionale, mediante l'approvazione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 42 del 2009, secondo le procedure di collegamento tra Parlamento, Governo e autonomie, previste dalla legge medesima. Diventa dunque un obiettivo irrinunciabile e sempre più cogente. Sarà da avviare anche una graduale riduzione della pressione fiscale. La riduzione sostanziale della pressione fiscale è strettamente collegata ad una riduzione più drastica della spesa pubblica (come dicevo prima), necessaria anche per favorire il cambiamento dell'apparato pubblico in senso federale, che in fase di transizione deve consentire una diversa ripartizione della pressione fiscale dallo Stato agli enti locali e territoriali, senza comportare un aggravio non sostenibile per il contribuente finale. Va continuata la lotta contro il lavoro irregolare per favorire l'occupazione dei giovani. A nostro avviso, legando anche le problematiche, di cui parlavo prima, sulla bilancia commerciale e sul picco che esiste di importazioni e questa flessione o comunque una crescita omogenea delle esportazioni, dovremo continuare ad impegnarci nella tutela del *made in Italy* in tutte le sue declinazioni, dal tessile all'agroalimentare, e reclamare una maggiore tutela da parte dell'UE per la via europea al «fare impresa» nel rispetto dei lavoratori, dell'ambiente, della sicurezza, della salute, adottando adeguate misure di contrasto della concorrenza sleale di coloro i quali, nella produzione, nel commercio e nella finanza, non rispettano gli stessi valori.

scenari di documenti in chiave europea interpreti bene le necessità e i bisogni del nostro Paese e ci possa consentire di guardare con serenità e tranquillità al nostro futuro, se effettivamente accelereremo il processo sul federalismo.

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, è difficile prendere sul serio questa discussione su un documento che - come ricordava il relatore di minoranza all'inizio del nostro dibattito presenta come essenziale elemento di novità il fatto che sia «sostanzialmente e politicamente superato» (citando testualmente da pagina 3 del documento stesso), però facciamo finta di prendere sul serio il documento e cogliamo l'occasione per parlare della politica economica di questo Governo. Ahimè, parliamo del nulla e infatti il documento e i suoi allegati non sono altro che la fotografia - mi sembra - del passato, con un po' di presente e praticamente nulla sul futuro. Da questo punto di vista è un'ottima fotografia del suo estensore, il ministro Tremonti, che in questi anni nulla ha fatto per il futuro del Paese; nulla per una politica economica di sostegno all'innovazione e a quel tessuto di piccole e medie imprese che tanto faticosamente sta sta tenendo a galla l'Italia e che sarebbe anche in grado di reggere la sfida della globalizzazione se alle sue spalle sentisse il sostegno di un sistema, sostegno di cui invece non c'è stata traccia nelle politiche concrete di questo Governo e che non si riesce a trovare nemmeno tra le righe di questo inutile documento, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua natura; nulla per affrontare la drammatica crisi del lavoro, una crisi i cui effetti drammatici sull'occupazione ho l'impressione che ancora non li abbiamo visti e che sembrano non preoccupare il Governo che tutt'al più, con il suo Ministro del lavoro (del non lavoro, verrebbe da dire con una battuta), sembra impegnato a dividere i sindacati nella sua ossessiva ricerca dello scontro. in tutto il mondo l'intreccio della crisi economico-finanziaria con quella climatica e ambientale è stato colto anche come un'occasione per puntare sulla *green economy* quale una delle chiavi principali per costruire un futuro migliore; qui nulla. Troppo recente è il tentativo di affossare gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili che il ministro Tremonti ha provato a portare a termine con l'ultima finanziaria per doverci ritornare in questa sede nel dettaglio. incomprensibile, non solo per noi del Partito Democratico, ma anche per gli artigiani, per le imprese e per i cittadini, l'ostinato rifiuto del Governo di prorogare e di rendere stabile lo sconto fiscale del 55 per cento per le ristrutturazioni edilizie che prevedano misure di efficienza energetica. Si tratta di una misura introdotta dal Governo Prodi - lo voglio ricordare - che è stata già utilizzata da oltre 600.000 famiglie e che ha messo in circolo 12 miliardi di euro, in un settore, quale quello dell'edilizia, che è tra i più colpiti dalla crisi, e che ha permesso un risparmio consistente di energia e conseguentemente di emissioni inquinanti. Sembra inoltre che vi apprestiate a decidere un'ulteriore proroga per l'entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei sacchetti di plastica che non siano biodegradabili, una misura che avevamo previsto nella finanziaria del 2007 e che sarebbe dovuta entrare in vigore già il 1° gennaio 2010. Si tratta di una norma che premierebbe l'industria chimica più innovativa, quella che sulla sostenibilità e sul suo rapporto con l'agricoltura basa il suo sviluppo, l'unica in grado di assicurare il futuro a un settore che ha fatto grande nei decenni scorsi questo Paese e che oggi è davvero a rischio: si veda, a questo proposito, la vicenda istruttiva del polo chimico ternano. Sono solo tre esempi negativi, ma quello che manca completamente è un approccio in positivo, quello che è al centro delle proposte del presidente Obama negli Stati Uniti d'America, ma persino di Governi europei con cui condividete la stessa ispirazione politica - penso alla cancelliera Merkel in Germania o al primo ministro Cameron nel Regno Unito - ma non evidentemente la stessa visone di futuro. Voi rimanete saldamente agganciati al passato e anche questo documento lo prova.

non c'è nulla di nuovo, ad eccezione di un'opera che sarebbe davvero utile per il Sud, ovvero l'asse ferroviario Napoli-Bari, per il quale però, guarda caso, non sono previste risorse. Per il resto, si tratta delle solite infrastrutture cosiddette strategiche, sempre annunciate in ogni DPEF, ma mai realizzate.

Per anni ci avete detto che quell'opera non sarebbe stata a carico della collettività, del bilancio pubblico, forse per convincere i vostri alleati di maggioranza della Lega Nord dell'utilità dell'opera stessa.

di quanto questo documento e tutta intera la politica economica di questo Governo siano fatti di proclami

legge che la Decisione di finanza pubblica è atto sostanzialmente e politicamente superato. Questa espressione mi ha incuriosito; ho pensato e ho capito che in fondo si è trattato di un conflitto temporale tra documenti di finanza pubblica nazionale e documenti di finanza pubblica europea. Non si sarebbe usata questa espressione se la congiuntura che ha determinato il Governo alla presentazione del documento di manovra, con il relativo decreto-legge, nel non ci fosse stata, perché in quel caso, evidentemente, l'oggetto e la materia contenuti in quel decreto-legge sarebbero stati presenti in questo documento, onorevole Vice Ministro: mi sembra di aver capito sufficientemente bene che così sono andate le cose. Quindi, non è che ci si sia dimenticati della necessità di rendere al Parlamento un documento. Il fatto è - ripeto - che la congiuntura ha fatto sì che il contenuto di questo documento lo si trovasse in quello. Tuttavia questo non è un documento inutile, perché vi troviamo un inventario completo, preciso, puntuale e aggiornato che ci mette nelle condizioni di argomentare, così come stiamo facendo e come faranno i nostri colleghi oggi e domani, per dare al Governo la possibilità di preordinare il contenuto dei documenti richiesti

Governo, siamo preoccupati quanto voi della monumentalità del debito pubblico e siamo preoccupati se un giorno, per cause indipendenti dalla nostra volontà, il costo di esercizio dello stesso dovesse raggiungere dimensioni tali che il Paese non fosse in grado di sopportare. Allora, dobbiamo fare presto e bene. E in costanza di una realtà nazionale e sovranazionale che ci impedisce di far lievitare il prodotto interno lordo e di aumentare il gettito tributario, che solo in condizioni normali può consentire di ripianare o di ridurre il debito, pensiamo con insistenza e con interesse all'utilizzazione proficua dei fondi strutturali. Mi riferisco a quei fondi che oggi ci capita di utilizzare anche per gli ammortizzatori sociali, ma che riteniamo debbano essere utilizzati anche grazie alla delega che recentemente il Governo ha dato al ministro Fitto, per perseguire obiettivi di costruzione delle infrastrutture e di riequilibrio territoriale. Perché le infrastrutture sono la via che consente alle aree meno dotate del Paese, in un certo momento storico, di potersi riequilibrare e al fine di

l'impegno, affinché la risoluzione da sottoporre all'Assemblea contenga un'indicazione chiara e precisa su un settore di intervento che potrà entrare a far parte integrante dei documenti programmatici che il Governo deve presentare in sede europea. In particolare, essa riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali per la rivitalizzazione dei centri storici dei piccoli Comuni, prima del Meridione e poi del resto del Paese, in analogia con quanto si è fatto con i piani Urban per le grandi città, che hanno già dato i loro risultati. La legge sulla casa, per la vischiosità della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, non ha dato i risultati sperati, ma se il Governo si muoverà nella direzione di finanziare quelle opere, le chiedo espressamente di esaminare l'opportunità di adottare una risoluzione che vada in questa direzione. Si tratta di borghi e centri storici, sia rivieraschi che di zone interne, la cui rivitalizzazione avrebbe notevoli effetti positivi su una pluralità di ambiti: il commercio, il turismo, la tutela del territorio, la salvaguardia di elementi ambientali in contesti di particolare pregio. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Ne avrebbero giovamento l'occupazione e l'intera filiera produttiva edilizia, che oggi versa in condizioni critiche. Il primo obiettivo dovrebbero essere immobili di Comuni e borghi ubicati nel Mezzogiorno. Si tratta di individuare, inoltre, procedure semplici e immediate, con controlli rigorosi: il beneficio andrebbe indirizzato a proprietari privati di immobili, e quindi sarebbe da escludere il meccanismo del credito d'imposta, così da realizzare un vero e proprio villaggio turistico in ogni centro urbano d'Italia.

vero, infatti, che dobbiamo parlare dei documenti; ma fuori da quest'Aula ci sono coloro che lavorano tutti i giorni e che si potrebbero chiedere cosa facciamo perché questo cavallo, che ha mani e piedi legati e che si chiama popolo...

in Europa e nel mondo. L'Europa si sta interrogando a fondo su come cambiare, non i dettagli delle proprie carte, ma l'impianto del proprio patto di convivenza, mettendo al primo posto l'occupazione, con degli obiettivi ambiziosi. Questo è un primo punto che vorrei sottolineare, per richiamare l'attenzione. Si continuano a indicare dei dati falsamente rassicuranti. Immaginate

centinaia di migliaia di persone che escono dal mercato del lavoro: quindi non basta dire che abbiamo una disoccupazione ufficiale meno grave di altri. Un dato che colpisce, e che vorrei venisse messo in queste carte,

di occupazione che si potranno raggiungere non si vedranno prima di sei o sette anni, come media. È necessario intervenire per rovesciare l'inanità che traspare dalle pagine del documento, altro che questa lontananza! Questo è un punto di cui ci preoccupiamo tutti. Il tavolo delle parti sociali, che faticosamente sta discutendo per cercare di dare un contributo, parla proprio di come intervenire sui meccanismi della crescita, di cui l'occupazione è un punto fondamentale. Morando, hanno indicato a lungo quali sono le proposte concrete che si possono fare, anche gradualmente;

e di occupazione assolutamente prive di qualsiasi riflessione critica, è veramente di disarmante disonestà. Per quanto ci riguarda, speriamo davvero che fra 10-15 anni, quando sarà ampiamente superato questo Governo, si potrà rimettere in fila

prospettive pensionistiche allarmanti. Credo che sarebbe bene che il Governo, pur nella sua confusione, sentisse questi drammi.

come ho avuto occasione di affermare qualche giorno fa in Commissione lavoro, il documento che oggi viene portato all'attenzione dell'Aula è tardivo, perché redatto in ritardo rispetto a quanto previsto dalla stessa legge di contabilità, e praticamente privo di particolare significato, ricalcando quanto già stabilito con la manovra economica di luglio. Ci si limita a fare una fotografia della grave situazione dell'economia italiana. Non si prevede alcuno strumento per far fronte alla situazione attuale ed in particolare non si imposta, e neppure si abbozza, alcuna politica sociale di lungo periodo. Ancora una volta, insomma, si naviga a vista. Uno dei dati principali contenuti nella Decisione di finanza pubblica è quello relativo alla situazione del lavoro. Il tasso di disoccupazione si attesterebbe all'8,7 per cento nel 2010, con un aumento di circa 1 punto percentuale rispetto al 7,8 per cento La stessa percentuale sarebbe prevista nel 2011, mentre nel 2012 vi sarebbe una leggera flessione all'8,6 per cento. Tra luglio 2008 e luglio 2010 sono stati persi almeno 881.000 posti di lavoro. Impressionante, inoltre, il dato della disoccupazione giovanile. Le assunzioni sono in netto calo e i licenziamenti sono stati contenuti grazie al ricorso massiccio alla cassa integrazione. Per i prossimi anni si prevedono livelli occupazionali complessivi di gran lunga inferiori a quelli precrisi. Dunque, dalla gestione della crisi d'impresa con la cassa integrazione si dovrà necessariamente passare alla gestione della disoccupazione, con il concreto rischio che sia una disoccupazione di lungo periodo e che coinvolga migliaia di lavoratori. Secondo le recentissime stime del Centro studi di Confindustria del settembre 2010, l'andamento del reddito *pro capite* in Italia continua ad essere negativo. La crisi ha aggravato ulteriormente questo andamento al punto che il Paese sarebbe tornato ai livelli addirittura del 1998. Quella descritta nel rapporto di autunno dello stesso Centro studi è un'Italia più povera in assoluto, e ancor più in rapporto agli altri Paesi avanzati. Rinnovando l'allarme per il ritardo nelle riforme, il rapporto sottolinea, tra le questioni cruciali sul fronte dei ritardi per la modernizzazione, tre punti in particolare: la semplicità e la chiarezza delle regole per le imprese che, tuttavia, mi si permetta una valutazione personale, non può e non deve tradursi, come sta avvenendo con il disegno di legge sulla semplificazione, nella semplice abrogazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il secondo punto è il carico fiscale sulle imprese e sui lavoratori; infine, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, terreno sul quale l'Italia è in forte svantaggio. Il Centro studi di Confindustria rileva che il ricorso alla cassa integrazione resterà alto per il resto del 2010 e che sono 450.000 i posti di lavoro persi a fine giugno, mentre altri 30.000 sono a rischio nella seconda metà dell'anno. Per Confindustria, insomma, il tasso di disoccupazione è ancora destinato a salire, terminando nel 2011 al 9,3

Dall'inizio della crisi al secondo trimestre 2010 sarebbero stati persi complessivamente nel nostro Paese oltre un milione di posti di lavoro. Colpiti per primi, come sempre, i lavoratori temporanei. Nella fase di picco della crisi, dei 508.000 posti di lavoro persi, circa 220.000 erano a tempo determinato. Le lavoratrici e i lavoratori attualmente in cassa integrazione sono oltre un milione e 200.000. Se si considerano tra gli inoccupati anche gli scoraggiati (circa 300.000 nuovi inattivi, soprattutto al Sud), il tasso di disoccupazione reale arriva all'11 per cento; e al 12 per cento con i lavoratori in cassa integrazione. Le imprese attualmente in stato di crisi sono oltre 5.000. Oltre 180 sono i tavoli di trattativa aperti per oltre 400.000 lavoratori. A tal proposito, non si può non sottolineare ancora una volta che questa gravissima situazione è stata affrontata male o in modo frammentario. Come è noto, il Governo si è permesso (ancora una volta per meri calcoli di tornaconto personale del Presidente del Consiglio) di lasciare senza titolare per ben sei mesi il Ministero dello sviluppo economico. Dal canto suo, il Ministro del lavoro ha ancora una volta preferito puntare sulla linea tutta ideologica della divisione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, degli accordi separati e dell'aggiramento normativo delle garanzie dei lavoratori. Il risultato di questo *mix* tra crisi e mancanza di efficaci azioni di rimedio è che il tasso di disoccupazione reale si prevede tornerà ai livelli precedenti la crisi solo nel 2017. L'ISTAT ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2010 è salito al 9,1 per cento (senza calcolare i lavoratori in cassa integrazione). Il dato più impressionante tuttavia resta, come accennato all'inizio, quello sulla disoccupazione giovanile. In Italia, secondo il CNEL, nel 2009 sono stati oltre 450.000 i posti di lavoro persi da parte dei giovani compresi tra i 16 e i 24 anni. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il picco del 28,2 per cento a febbraio 2010 e nel secondo trimestre si è attestata al 27,9 La media europea nell'anno 2009 è stata del 19,8 per cento. Nel Mezzogiorno l'indice arriva addirittura al 39,3 Secondo l'ISTAT, nel 2009 il numero dei giovani che non lavorano e non frequentano nessun corso di studio o di formazione superava di poco i due milioni: rappresentano il 21,2 per cento della popolazione tra i 15 e i 29 anni. Per quanto riguarda coloro che hanno - per loro fortuna - un impiego, il 30 per cento della popolazione tra i 18 e i 29 anni svolge un lavoro atipico. Come già precisato, è proprio in tale segmento che si è concentrato il calo maggiore dell'occupazione. Sempre secondo l'ISTAT, se per ogni 100 giovani occupati nel primo trimestre 2009, a distanza di un anno, 15 sono transitati nella condizione di non occupato, tra i giovani con contratto di collaborazione questa percentuale sale a 27. Cresce inoltre la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza. Secondo l'ultima indagine di Banca d'Italia sui redditi delle famiglie italiane, il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede quasi il 45 per cento dell'intera ricchezza netta delle famiglie italiane.

11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171 euro. La distanza tra la ricchezza netta media (137.956 euro) e la ricchezza netta mediana di quel 50 per cento più povero (cioè 68.171 68.171 euro), evidenzia in maniera lampante l'iniquità della distribuzione. Nel 2008, i redditi maggiormente dichiarati al fisco sono stati quelli da lavoro dipendente e da pensione, sia in termini dì frequenza (86 per cento) che di ammontare (78

per cento dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l'anno e il 40,04 per cento dichiara redditi tra 15.000 e 35.000 euro. E solo lo 0,9 per cento dei contribuenti dichiara redditi superiori ai 100.000 euro annui. In totale, il 90,90 per cento (oltre 37 milioni di contribuenti) dichiara meno di 35.000 euro. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti è pari a 19.280 euro.

incontestabile situazione, emerge invece come prioritaria ed urgente la necessità di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro, sulle pensioni e sugli investimenti delle piccole e medie

L'unica alternativa possibile alle scelte sbagliate di questo Governo è una politica di sviluppo: l'impegno serio e responsabile di maggiori risorse

Signor Presidente, ciò che immediatamente colpisce della Decisione di finanza pubblica è l'affermazione del Governo secondo cui tale documento è già «sostanzialmente e politicamente superato», perché quanto doveva essere deciso è già stato fissato nel luglio scorso e perché la discussione di politica economica sarà all'interno del nuovo schema europeo. È dunque il Governo a deprezzare in premessa la Decisione di finanza pubblica come documento di programmazione economica e finanziaria. Il Partito Democratico non accetta questo *a priori*; non accetta la svalutazione sistematica che questo Governo fa del Parlamento e della necessità che Camera e Senato concorrano al processo decisionale di programmazione economica e finanziaria con il necessario rispetto politico, oltre che istituzionale, e per i tempi e modi di approfondimento ed elaborazione. Non accettiamo inoltre che il vincolo europeo, e soprattutto lo spirito della nuova strategia europea di coordinamento, che in realtà rappresenta l'inizio della nuova costituzione materiale, ma anche formale dell'Europa dopo la crisi finanziaria, anziché essere considerato per un Paese come l'Italia una straordinaria opportunità, a fronte delle sue criticità strutturali, venga utilizzato come alibi e come tentativo di sterilizzare questo passaggio da ogni implicazione politica e strategica. Voglio dare atto alla relatrice, senatrice Bonfrisco - non era facile, ha fatto veramente per questo una relazione onesta - di aver voluto ricordare in premessa

agli obiettivi programmatici dei saldi per il complesso delle pubbliche amministrazioni. Ma la portata di queste implicazioni viene poi di fatto azzerata, si è detto era necessario soprassedere e cioè piegare la pianificazione strategica nazionale al nuovo modello europeo. Le cose non possono essere poste in questi termini. Se è ovvio che la modifica delle regole europee comporterà modifiche per tutti, è altrettanto evidente che, nella fase transitoria, la bozza del Piano nazionale di riforma che gli Stati membri dovranno presentare entro il 12 novembre prossimo poteva trovare in questo *step* parlamentare l'occasione per mettere a punto l'analisi degli squilibri, l'identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento della occupazione e le misure strategiche di riforma da adottare per perseguire obiettivi di crescita finanziaria e occupazionale. È proprio questo che, una volta di più, non si vuole fare in questo Parlamento. In questi anni tanto difficili per l'Italia, e anche per l'Europa nel mondo globalizzato, questo Governo si assume la responsabilità di non fare la cosa giusta, quella di rivolgersi alle energie migliori del Paese, unire gli sforzi, chiamare alla responsabilità e alla solidarietà verso chi nella crisi paga il prezzo più alto, né fare quella necessaria: rivolgersi a tutto il Parlamento e chiedere lo sforzo più alto di responsabilità. L'Europa, dunque, intesa come pretesto per dilazionare e non come opportunità e stimolo per reagire e superare lo stallo e l'inerzia in cui versa il sistema Italia. In Europa, invece, non va così: la crisi finanziaria con le ricadute sull'economia reale e sull'occupazione è stata piuttosto l'occasione per portare alla luce e porre rimedio ad una pericolosa lacuna del processo di integrazione europeo, e cioè il mancato equilibrio tra le misure monetarie sopranazionali centrate sull'euro e le politiche economiche nazionali insufficientemente coordinate. È in questo contesto e in un frangente critico come l'attuale che si è visto come il persistere di un tale squilibrio avrebbe minacciato la stessa Unione monetaria e compromesso la prospettive di stabilità dell'euro. Raggiunta la consapevolezza che in Europa la crisi, con tutte le sue implicazioni sia di instabilità finanziaria che di ricaduta sulle imprese e sull'occupazione, sarebbe stata aggravata da politiche di bilancio scorrette dei Paesi membri e, anche grazie alla severità della BCE, è stato disinnescato l'attacco contro il debito sovrano della Grecia, dimostrando così anche la capacità dell'Unione europea di fronteggiare altri eventuali attacchi ai debiti sovrani della zona euro. Una decisone determinata che ha fatto giustizia anche di tante previsioni fosche sul crollo dell'euro e dunque del fallimento dell'Unione. Di qui la straordinaria evoluzione in corso e la prospettiva concreta di una *governance* europea dell'economia, fino all'assoluta novità comunitaria dell'iniziativa congiunta dei due leader, francese e tedesco, in vista addirittura - si parla - di una convergenza dei sistemi fiscali di Francia e Germania. In questo quadro di iniziative, impensabili solo un anno fa, in Europa sta maturando la nuova *governance* europea a cui Francia e Germania vorrebbero dare una forte valenza politica. Per il futuro, dunque, le decisioni nazionali di finanza pubblica, come le politiche di bilancio, le politiche macroeconomiche e le riforme strutturali saranno prese a livello comunitario, tenendo conto delle diverse situazioni dei Paesi membri. La domanda che vorrei porre è se il Governo pensa che il nostro Paese possa concorrere, e come, a questo nuovo processo regolativo o se, viceversa, dobbiamo considerare che, date le nostre condizioni di salute, e in particolare di debito, non possiamo che assistere passivamente e sperare che il nostro dolce far niente possa di per sé salvaguardarci. In Europa si discute di regole: regole per la finanza, ma anche regole per l'economia. Ritorna in tutto il mondo il tema del governo dell'economia, e noi cosa ne pensiamo Non vi è nemmeno traccia in questo schema di DFP delle cinque priorità messe dal Governo al centro del programma su cui è stata chiesta la fiducia al Parlamento solo una settimana fa. E tra queste, ancora una volta, non vi è traccia né menzione di quel Mezzogiorno che più di ogni altro territorio dell'Italia ha sofferto la mancanza di crescita e di politiche efficaci per la crescita. Da tempo abbiamo smesso di fare politiche industriali. E cioè abbiamo smesso da tempo di chiederci: cosa deve fare il mio Paese, la mia Regione? Verso quali vocazioni dobbiamo orientarci? Abbiamo tutti, certo - non solo gli italiani - più o meno teorizzato che l'unica politica industriale fosse quella della concorrenza (salvo poi, noi, non curarci nemmeno di quella). E una volta finiti i sussidi, che hanno rappresentato la forma italiana di politica industriale di cui hanno beneficiato le imprese numero uno (o presunte tali, come l'Alitalia per ultima), c'è stata una paralisi totale. Sono persuasa che la posizione italiana in Europa sarebbe più forte se, insieme al rigore dei conti, ci presentassimo con un profilo riconoscibile nel merito di scelte non più rinviabili per il Paese. Non voglio soffermarmi nel merito delle nostre proposte, qui illustrate ampiamente dal senatore Morando; vorrei, invece, insistere su un punto. Certamente possiamo essere più credibili in Europa se il nostro Paese, tanto deluso, si dimostrerà e si percepirà come un Paese capace di recuperare la delusione e ritrovare le ragioni di una fiducia in una prospettiva. Ma la cosa più drammatica in questo questa prospettiva non ci viene indicata; proprio per questo si naviga a vista. Questo documento è il sintomo eloquente di una inerzia che non solo viene praticata, ma che addirittura si pretende di predicare. Una inerzia inaccettabile e politicamente preoccupante nei confronti dell'economia, del Paese reale, della sofferenza di tante famiglie e di tante persone, sopratutto giovani, che non vedono più un futuro. Tutti i dati di cui disponiamo, in definitiva, ci parlano proprio dell'inerzia che caratterizza il presente e dell'impossibilità di vedere un futuro. Questo chiama in causa tutta la classe dirigente; *in primis* il Governo, che si ostina a proporre linee previsionali puntualmente smentite dai fatti, e poi l'opposizione, le cui proposte qui illustrate sono chiamate anch'esse alla prova della pubblica opinione. Una prova difficile, che chiama in causa l'intera *élite* del Paese in un passaggio tra i più stretti della storia repubblicana. Una prova che chiede il massimo di rigore e di serietà, ma anche di speranza e di fiducia nelle nostre possibilità, che sono reali. Vorrei citare due esempi: uno è il nostro sistema manifatturiero. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che dopo la Germania è l'Italia a mantenere un solido sistema manifatturiero, seppure concentrato solo al Centro-Nord, che in qualche modo rappresenta la nostra polizza assicurativa, con il suo patrimonio di competenze, di imprese e di lavoro, per un futuro di ripresa economica. Il secondo esempio riguarda il Mezzogiorno d'Italia, che è tanta parte del Paese, con i suoi straordinari giacimenti ambientali, culturali, artistici, con straordinarie potenzialità economiche, al contrario di ciò che pensa Tremonti quando dice che la cultura non si mangia. Non solo noi dobbiamo credere nella rinascita del Mezzogiorno, perché un Sud tanto arretrato non è più sostenibile per il Paese, ma possiamo crederci, se assumiamo una visione strategica di rottura dell'inerzia del presente, di cui ha bisogno l'Italia intera, e se favoriamo l'esplosione delle energie migliori, oggi compresse, innanzitutto facendo leva sul dinamismo dei giovani e sulla responsabilità delle donne. È soprattutto a loro che dobbiamo saper parlare ed è con loro che si può curare il presente e guardare al futuro. Non è quello che fa il Governo; non lo fa con la non-Decisione di finanza pubblica. Dal Governo, dunque, ora non c'è niente da aspettarsi a breve. C'è, però, molto da criticare, e noi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vice ministro Vegas, tralascio volutamente di commentare dal punto di vista tecnico e giuridico lo schema di Decisione di finanza pubblica, che, com'è noto, sostituisce il DPEF, Documento di programmazione economico-finanziaria. Rilevo solo che si agisce ormai alla luce della incipiente riforma della politica economica europea. La parte più importante del documento è l'analisi macroeconomica, un quadro di riferimento utile a prospettare le linee per la definitiva uscita dalla crisi: un'analisi seria e fondata - di cui diamo atto al ministro Tremonti - che mette in luce aspetti positivi, come la tenuta dei conti per la spesa pensionistica, ma che evidenzia anche le criticità, come il tasso di disoccupazione, che nel triennio considerato fatica a scendere, e la stagnazione dei consumi. Relativamente ai conti pubblici, le previsioni indicano un livello di indebitamento netto tendenziale in riduzione fino al 2,2 per cento Tale prospettiva è legata alla significativa riduzione delle spese complessive, un obiettivo ottenuto grazie alla decisa azione del Governo nella riqualificazione della spesa pubblica. Per quanto riguarda poi l'evoluzione del rapporto debito-PIL, l'atto conferma l'andamento discendente di tale rapporto. Il picco del 2011 è dovuto alle maggiori emissioni necessarie per finanziare i contributi italiani alla Grecia. Un aspetto altamente positivo che rilevo con soddisfazione si evince dall'analisi delle entrate tributarie, le quali nel periodo considerato registrano un incremento dello 0,5 per cento in rapporto al PIL, una crescita determinata quasi esclusivamente dalle norme in materia di lotta all'evasione fiscale e contributiva recentemente adottate. Non cresce quindi la pressione fiscale, che ha raggiunto nel 2009 il 43,2 per cento e dovrebbe nel triennio successivo attestarsi su un livello inferiore, toccando il 42,4 per cento nel 2013: di poco, ma cala. Prende corpo, pur in una situazione difficile caratterizzata da un alto deficit pubblico e da ingenti spese per gli ammortizzatori sociali, un impegno preso dal Governo: riforma fiscale è uno dei punti del programma: noi la aspettiamo e ci crediamo. Ci auguriamo dunque di realizzare questo obiettivo, addirittura prima della riforma prevista, come uno dei punti programmatici di coalizione. Dopo questo importante riconoscimento al Governo, voglio però dire che è necessaria una svolta nella politica economica. Occorre trovare le risorse per sostenere le imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro, perché c'è disoccupazione. Se, come è scritto, la ripresa economica mondiale si sta consolidando alcuni dati confermano che l'industria italiana si risveglia: la produzione segna un passo in avanti del 9,5 per cento rispetto ad un anno fa

Dopo i tonfi del 2009 e le incertezze di luglio, i risultati abbattono le previsioni e lanciano la locomotiva tricolore all'inseguimento della Germania, unico tra i Paesi europei che fa meglio di noi (mi dispiace, non condivido quanto è stato detto dalla sinistra). L'industria non si è data per vinta e ha ribaltato le previsioni, con buona pace - devo dire - di Montezemolo e grande soddisfazione - suppongo - di Emma Marcegaglia. Resta la necessità di sostenere la capacità di penetrazione italiana sui mercati internazionali, specie dove l'economia cresce di più. Occorre dare alle imprese le risposte che attendono, nel senso cioè di essere messe in condizione di intraprendere e di investire: solo così vinceremo la sfida per mantenere l'Italia tra gli otto grandi Paesi del mondo, Certe azioni dell'Esecutivo, di cui ho ricordato alcuni importanti risultati, vanno senza dubbio in questa direzione: penso allo snellimento burocratico, all'aumento dell'efficienza dello Stato, Stato, alla riforma scolastica, alla politica internazionale (sono solo pochi di possibili esempi). Il Governo è andato bene. Sarebbe però una sconfitta per tutti se esso, in relazione alla disciplina del Patto di e al rafforzamento della *governance* economica dell'Unione, fosse bloccato nel suo agire dal pur condivisibile obiettivo di garantire stabilità di lungo periodo nelle politiche di bilancio. L'Unione europea non svolgerebbe bene il proprio ruolo se privasse i Governi nazionali degli strumenti di politica economica indispensabili per sostenere la crescita, rilanciare gli investimenti e la ricerca e migliorare il livello di competività dell'economia. Occorre riproporre con più convinzione a livello nazionale un'impostazione di politica economica che, garantito l'equilibrio di bilancio, liberi risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali. Ciò sarà possibile riequilibrando il carico tributario a favore del lavoro, per esempio, dei fattori produttivi dell'economia reale e sostenendo una maggiore capitalizzazione delle imprese. Ho già chiesto al Governo di attivarsi a livello internazionale per dare nuove e condivise regole ai mercati finanziari, per rafforzare i meccanismi a garanzia dell'adeguatezza patrimoniale delle banche, a fronte dei finanziamenti da esse erogati, in modo che non si determinino ricadute negative sulla effettiva disponibilità di credito al sistema produttivo, in particolare, alle piccole e medie imprese. Anche il completamento della riforma in senso federalista del sistema tributario dovrà ispirarsi al principio di responsabilità di bilancio e di orientamento alla crescita dello strumento tributario, assicurando un maggiore coinvolgimento di tutti i livelli di governo nelle scelte fondamentali di politica economica. Mi auguro che questi aspetti di programmazione vengano considerati nel Piano nazionale di riforme che sarà la logica prosecuzione di questo schema di Decisione di finanza pubblica. Nel manifestare il mio voto favorevole, so di impegnare il Governo a questa azione di rilancio economico azione di rilancio economico con quella capacità innovativa nelle soluzioni che ha sempre contraddistinto il Presidente del Consiglio e, lasciatemelo dire, il mondo imprenditoriale italiano, che è in grado di farlo. *(Applausi

Signor Presidente, signor Vice Ministro, purtroppo stiamo esaminando un documento privo di contenuti significativi, elusivo e rinunciatario. Dallo schema di Decisione di finanza pubblica emerge plasticamente la conferma di una risposta debole da parte del Governo e della maggioranza, del tutto inadeguata rispetto alle criticità e alle aspettative della realtà sociale e produttiva del Paese, segnata pesantemente dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria e più che mai bisognosa di interventi a sostegno della competitività, dell'occupazione, dei redditi dei lavoratori e delle famiglie. Ben lungi dalle rassicurazioni sul fatto che i conti sono in equilibrio e che «tutti gli interventi necessari sono già stati assunti», così da rendere di portata minimale la imminente sessione di bilancio, le audizioni svolte nelle Commissioni competenti di Camera e Senato hanno invece chiaramente che per il nostro Paese la situazione competitiva non è per nulla rassicurante e pretendono piuttosto, quelle sollecitazioni venute, che dal lato della finanza pubblica si metta mano velocemente a misure sostanziali e di significativa portata. È evidente che sulla operatività del Governo pesano i problemi interni alla maggioranza, e questo basso profilo risulta clamorosamente ancor di più per la completa omissione di coerenza rispetto ai cinque punti su cui solo dieci giorni fa il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia delle Camere. In particolare, sul punto della riforma fiscale, definita ancora una volta dal Presidente del Consiglio «una chiave strategica per la crescita del Paese» con la reiterazione della promessa (ormai divenuta un po' stucchevole) di ridurre la pressione fiscale, «tenendo conto - cito le sue parole - delle esigenze e delle compatibilità di bilancio pubblico, sulla base della lotta all'evasione fiscale e del dividendo della crescita». Come a dire: vorrei ma non posso, quindi mettetevi il cuore in pace. Infatti, l'obiettivo non è compatibile con i numeri forniti nella Decisione di finanza pubblica di cui oggi discutiamo, che, invece, prevede la pressione tributaria in aumento di 0,3 punti percentuali, nonostante il venir meno di 0,8 punti di gettito conseguenti allo scudo fiscale e ad altri interventi straordinari. Sembrerebbe, dunque - ed è già stato sottolineato - che il prospettato recupero dell'evasione, insieme all'auspicato dividendo della crescita, si tradurrà di fatto in un aumento delle imposte. Né si evince, dal documento di finanza pubblica, come potrà concretizzarsi una riduzione graduale del prelievo su famiglie e imprese in coerenza con l'evocazione, fatta sempre dal Presidente del Consiglio nell'illustrazione delle cinque priorità di azione del Governo, del quoziente familiare (uno slogan, nulla più) e del taglio dell'IRAP, scaricato interamente sulle spalle delle Regioni a cui, contemporaneamente, sono state drasticamente ridotte le risorse. Su questi temi, invece, bisognerebbe aprire un confronto serio, perché a nessuno sfugge che la tenaglia entro cui è stretta la finanza pubblica del nostro Paese condiziona e limita gli spazi di intervento. La possibilità di ridurre il prelievo fiscale è realisticamente legata ad un effettivo recupero dell'evasione, che ha tuttavia, se perseguita con una strategia organica e continuativa, ampi margini per conseguire rilevanti risultati; così come un'azione fiscale che persegua obiettivi di maggiore equità ed efficienza può avvenire anche attraverso una redistribuzione del prelievo, e non solo attraverso una sua riduzione.

del lavoro dipendente o di pensione o che, comunque, si inseriscono negli spazi più bassi della scala sociale mettono in evidenza che oggi redistribuire è un'esigenza imprescindibile, non solo per ragioni di equità, ma anche per sostenere e contribuire a rilanciare i consumi. Certo, la sfida di una riforma su questi temi è estremamente complessa, ma non può essere più rinviata o elusa. La settimana scorsa, come è noto, all'Assemblea nazionale tenutasi a Varese, il Partito Democratico ha provato a sistematizzare le linee di un disegno complessivo ed organico di riforma, che ha come elementi caratterizzanti per la riallocazione del prelievo alcuni profili che cercherò sinteticamente di richiamare. Da chi paga a chi non paga, attraverso la lotta all'evasione e all'elusione, come già detto, e lavorando al meglio sia sulla *compliance* dei contribuenti, sia utilizzando l'accesso e l'incrocio delle banche dati consentiti dalle tecnologie. Dai redditi da lavoro alla rendita, per alleggerire il carico che oggi grava eccessivamente sui produttori di reddito da lavoro e d'impresa.

da premiare le responsabilità familiari, ma anche, considerando il problema dell'incapienza, prevedendo l'introduzione di un *bonus* per i figli e la previsione di consistenti agevolazioni fiscali a sostegno dell'occupazione femminile. Da attività inquinanti ad attività verdi, perché siamo convinti che la fiscalità può rappresentare una leva decisiva per sviluppare una *green economy* e orientare l'economia verso la sostenibilità ecologica (si tratta di temi su cui nel documento in discussione non c'è assolutamente traccia). Dalla dimensione nazionale al territorio, facendo del federalismo non un motivo di propaganda a buon mercato, ma una leva per un'effettiva modernizzazione del Paese, ponendo il tema della fiscalità e dell'autonomia impositiva delle istituzioni sul territorio in coerenza con una visione di riforma complessiva del sistema fiscale. Le due questioni infatti, sono interdipendenti e ignorarlo comporta dire trovarsi di fronte a decreti attuativi assimilabili a scatole vuote, senza numeri, con incertezza di garanzie sui livelli delle prestazioni e sulle funzioni fondamentali, oltre ad una mancanza di obiettivi certi di perequazione e sviluppo. Insomma, un *bluff*, che anche con le nostre proposte intendiamo smascherare. ricordare un insieme di proposte qualificanti ed innovative per una riforma del prelievo sui redditi di impresa e di lavoro autonomo, in primo luogo prevedendo di eliminare, gradualmente, l'IRAP sul costo del lavoro.

a partire dall'appuntamento di presentazione al confronto parlamentare e poi di discussione della legge di stabilità. Non perdiamo almeno quest'ennesima occasione, anche perché a fronte dell'urgenza di assicurare risposte sulle linee che ho richiamato,

che il Ministro dell'economia si presentasse al confronto parlamentare per valutare le priorità di destinazione di questo eventuale maggiore gettito, che non

a una detrazione fiscale specifica per le madri lavoratrici, al fine di contribuire alla copertura dei costi connessi agli impegni di cura e sostenere l'occupazione, e soprattutto la riduzione della pressione fiscale nei confronti dei percettori di reddito da lavoro e di pensione attraverso l'innalzamento delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché questa è una necessità di cui assolutamente il Paese ha bisogno e, in particolare, ne hanno bisogno quei lavoratori, quei pensionati.

partiamo da una premessa di metodo: la Decisione che stiamo esaminando è destinata ad essere superata alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Il suo contenuto programmatico, quindi, potrebbe essere oggetto di revisione nella prossima primavera, ma ciò non ci impedisce di fare alcune brevi annotazioni. Il quadro delineato dalla DFP ci fa intravedere uno scenario tra luci ed ombre. Tutto quanto fatto in questa legislatura finora ha consentito di raggiungere un obiettivo ineludibile: contenere il deficit entro limiti fisiologici per una fase di crisi dell'economia mondiale. La scelta del Governo di anticipare la manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013 con il decreto-legge n. 78 del 2010 per mantenere gli impegni assunti in sede europea ci ha consentito di sopportare meglio di quanto avvenuto in molti altri Stati gli effetti della crisi mondiale. È stata salvaguardata la stabilità finanziaria del Paese nonostante il grave vincolo costituito da un ammontare di debito pubblico particolarmente ingente. Noi riconosciamo pertanto la serietà dell'impegno con il quale è stato finora condotto il Paese in due anni difficili, segnati dalla peggiore crisi economica del dopoguerra, ma è evidente che ciò ormai non basta più. Non basta nei confronti di un Paese che si ritrova stanco, afflitto da problemi decennali che si sintetizzano in un solo dato: la più bassa crescita media dell'ultimo decennio tra i Paesi più sviluppati. Preoccupanti sono infatti i segnali di rallentamento emersi nel terzo trimestre di quest'anno. Le prospettive di crescita non risultano ancora stabili, come segnalato dalla DFP, la quale rivede infatti dall'1,5 per cento all'1,3 per cento il tasso di incremento del PIL nel 2011. All'interno di questo dato ci preoccupa poi l'andamento della disoccupazione reale, piuttosto che di quella cifrata dall'ISTAT. Difatti, se si è riusciti a contenere il tasso di disoccupazione in questi ultimi due anni ciò è dovuto anche all'ampio utilizzo della cassa integrazione in deroga. Su questo fronte sono state impegnate risorse ingenti, ma va anche ricordato che quelle stesse risorse sono state attinte, in massima parte, dal FAS (Fondo aree sottoutilizzate), che a sua volta, con il decreto-legge n. 185 del 2008, ha finanziato il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. La disoccupazione ormai è un problema nazionale e al Sud è emergenza. Al Sud, infatti, la disoccupazione reale si colloca, secondo alcuni, sopra il 20 per cento, di circa sei punti in più rispetto al dato ufficiale calcolato dall'ISTAT. Sono lavoratori scoraggiati; è evidente che una gran parte di queste persone è andata ad alimentare l'abusivismo, il lavoro nero e spesso anche la delinquenza. sosteniamo pertanto che il tema della bassa crescita della produttività debba essere posto al centro del dibattito di politica economica italiana. Riteniamo positivo dunque l'avvio del confronto tra imprese e organizzazioni sindacali, purché esso abbia un orizzonte ampio e di respiro lungo e non voglia invece limitarsi alla considerazione delle deroghe al contratto collettivo nazionale, ma ci preoccupa il fatto stesso che le parti sociali si siano avviate su questo cammino in parte prescindendo dall'atteggiamento del Governo, come se su questo fronte ci si sia rassegnati a dover fare da soli. È un sintomo preoccupante di un certo scollamento tra sistema produttivo e politica, che non va trascurato. indispensabile, sull'assoluta necessità di mantenere salda la linea del rigore finanziario in termini di controllo del deficit pubblico e, possibilmente, di ripiegamento - il più rapido possibile - del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Tutto ciò non toglie, però, che vi sono molti punti sui quali raccomandiamo maggiore incisività. Occorre passare dai proclami alle azioni concrete. L'azione di risanamento portata avanti fino ad oggi non ha affrontato i nodi strutturali della nostra finanza pubblica: il livello di evasione senza pari nell'ambito dell'Unione europea e la necessità di razionalizzare la spesa pubblica rendendola più efficiente. In Italia il livello di pressione sui redditi da lavoro dipendente, cresciuto nel tempo, è divenuto insostenibile. Nel breve periodo occorre una attenta verifica della sostenibilità del processo di federalismo fiscale: occorre incentivare una sempre maggiore partecipazione degli enti locali, specie dei Comuni, all'azione di efficientamento della spesa pubblica e del contrasto all'evasione. Occorre farlo non solo per incrementare il gettito erariale, ma soprattutto per realizzare una più equa ripartizione dell'imposizione tributaria e per reperire risorse aggiuntive senza incrementare la pressione fiscale sui contribuenti onesti. Solo così potremo impostare l'attuazione del quoziente familiare, l'introduzione della cedolare secca e tutte quelle riforme che avevamo promesso ai nostri elettori, e su cui ci siamo già spesi, presentando l'anno scorso un ordine del giorno accolto dal Governo.

è elevato. Nel medio periodo occorre fare scelte lungimiranti. Bisogna individuare quelle sacche di parassitismo e di spreco che ancora oggi esistono all'interno della spesa pubblica, passare dalla politica dei tagli orizzontali, che penalizzano tutti i settori dello Stato, a tagli verticali che individuino settori improduttivi e inutili, per investire laddove si ritiene opportuno, implementando gli interventi necessari in settori come l'educazione, la scuola e la ricerca: altrimenti, rischiamo di condannare il Paese all'impoverimento culturale e alla decadenza economica e sociale. fine del mese scorso, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che l'azione del Governo, in campo economico, si concentrerà sui temi del federalismo fiscale, della riforma tributaria e del Sud. Vi è ampio timore che a beneficiare del federalismo possano essere le aree meno sviluppate del Paese. Esiste poi il rischio di un federalismo «per abbandono», che incrementi e renda più complicata la gestione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. Dobbiamo evitare tutto questo, ma possiamo farlo solo se il processo non viene imposto a scatola chiusa: occorre aprire la scatola nera dei numeri del federalismo e vedere cosa c'è dentro, senza attendere gli anni che servono per la sua attuazione definitiva. Ricordo a tutti noi che anche il modello di federalismo fiscale attualmente vigente, quello concretizzatosi nel ben noto decreto legislativo n. 56 del 2000, ha patito una fase di arresto sostanziale, in quanto solo *a posteriori* le Regioni hanno compreso le sue ricadute finanziarie: esiste anche ora il rischio del ripetersi di un simile insuccesso. Soprattutto deve essere garantito quello che il Presidente del Consiglio ci ha promesso: poter usufruire di servizi pubblici di uguale livello e qualità in tutto il territorio nazionale. Mi avvio alla conclusione: il Sud continua ad essere un enorme serbatoio di risorse umane sottoutilizzate,

sottoutilizzate, è l'area del Paese che ha più margini di crescita, ma la gestione dei fondi FAS di questi due anni deve essere sicuramente rivista. Dobbiamo tornare allo spirito del 1994, realizzando quella rivoluzione liberale che prometteva meno tasse e meno spesa pubblica,

non intendo soffermarmi sui ritardi che hanno caratterizzato la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP), un documento programmatico nuovo, appena nato, ma praticamente già superato. Ci tengo però a dire che il rispetto del termine di presentazione di questo documento è un elemento fondamentale, poiché, quanto più in ritardo viene presentato, tanto più improbabile diviene la possibilità di recepire le indicazioni parlamentari. Questo documento riflette solo decisioni già prese, praticamente inconsistenti, così come inconsistente è il contenuto dell'Allegato infrastrutture, relativamente al quale, prima di entrare nel merito, è opportuno ricordare che la trasmissione del documento è avvenuta dopo la comunicazione agli organi di stampa. Si è scelto, cioè, di dare precedenza al «Sole 24 ore» piuttosto che alle Camere. Il quotidiano pubblicava infatti, il 5 ottobre scorso, un articolo riportante la sintesi dettagliata delle 28 priorità infrastrutturali individuate dal Governo. A questo punto, forse, dobbiamo dedurre che il messaggio che volete darci è che dobbiamo rassegnarci e assistere impotenti al ripetersi di atteggiamenti di sgarbo nei confronti delle istituzioni. Ma veniamo al contenuto dell'Allegato. La prima considerazione che mi viene da fare è se, alla luce del suo contenuto, questo documento possa ancora essere considerato utile. La natura confusa che lo contraddistingue è frutto di un'elaborazione approssimativa, con cifre che vengono riportate in modo, ahimè, inesatto. A ciò occorre aggiungere che il documento viene redatto ogni anno secondo metodologie diverse, rendendo quindi difficile, e forse inutile, ogni tipo di confronto sui dati, confronto però necessario per poter avere il quadro completo dello stato di avanzamento dei lavori. Ci è stato presentato - come ho detto - un provvedimento che fa dubitare fortemente della centralità che il Governo Berlusconi dichiara di riconoscere alle infrastrutture; un settore nel quale, sin dall'approvazione nel dicembre 2001 della legge obiettivo, il Governo di allora, così come quello attuale, hanno puntato su operazioni di finanza creativa, che non hanno consentito di conseguire i risultati sperati, a fronte anche del cattivo andamento dei conti pubblici. Non è un dettaglio il fatto che uno dei maggiori difetti del programma delle infrastrutture strategiche sia il suo gigantismo rispetto alla limitatezza delle risorse pubbliche disponibili. Nel campo delle infrastrutture, l'indifferenza al principio di realtà e il rigetto così radicale del metodo della programmazione non hanno eguali. In questi dieci anni, la scarsità delle risorse economico-finanziarie non è stata neppure lontanamente considerata come condizione necessaria per procedere davvero ad una selezione delle opere effettivamente necessarie. Il numero di opere strategiche è variato notevolmente nel tempo, passando dalle 88 stimate nel 2001 alle 348 cui si riferisce il V Rapporto, aggiornato al 30 aprile 2010,

A fronte di tali dati, il quadro che emerge dall'Allegato infrastrutture, che dovrebbe essere, signor Vice Ministro, un documento informativo chiave in ambito infrastrutturale, non è per nulla chiaro quanto a trasparenza dei dati relativi alle risorse disponibili, né tanto meno rispetto alle priorità degli interventi. È singolare che l'importo delle opere del programma sia riportato senza indicare l'ammontare puntuale delle risorse destinate ad ogni singola opera e, soprattutto, che il valore non coincida affatto con quello indicato dal V Rapporto sullo stato di attuazione della legge obiettivo, i cui dati recentissimi risalgono - ripeto - al 30 aprile 2010. Il documento definisce fisiologico il passaggio da un costo di 126 miliardi del 2001 ai 231 miliardi del 2010; peccato che non sia chiaro quale dato bisogna ritenere reale: quello del Governo o quello del Rapporto?

per recuperare il *gap* infrastrutturale che penalizza il nostro Paese nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea. L'Italia è un Paese in crisi, ma la crisi economico‑finanziaria che l'ha investita nell'ultimo biennio non relega in secondo piano il problema delle infrastrutture. Al contrario, tra i principali strumenti per superare la recessione e rilanciare la crescita vi è notoriamente la realizzazione di grandi programmi pubblici di sviluppo e ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture strategiche. Non a caso, importanti investimenti di lungo periodo in infrastrutture nel settore dei trasporti, dell'ambiente, della produzione e distribuzione di energia e dell'infrastrutturazione urbana rappresentano una componente fondamentale delle strategie dei diversi tra i maggiori Paesi. Il Presidente degli Stati Uniti, proprio poche settimane fa, ha deciso di investire 50 miliardi di dollari sulle infrastrutture e sui trasporti, nella consapevolezza che da questi settori passa il rilancio dell'economia e dell'occupazione, quindi della ripresa. Dovrebbero essere questi i terreni privilegiati di un confronto politico condotto con impegno e con l'intento di trovare soluzioni largamente condivise, dunque di giungere a trovare rapidamente Non serve il muro contro muro, non serve continuare a raccontare favole sulle cifre, sui dati, su quanto si è fatto e si deve ancora fare: bisogna iniziare a lavorare sul serio. In un documento di pianificazione, il Governo dovrebbe essere chiamato a mettere nero su bianco, in maniera oggettiva, ciò che ha fatto e ciò che intende fare. L'Allegato infrastrutture non può ridursi ad essere la fiera dei propositi e delle buone intenzioni. Si giunge addirittura a parlare di un piano strategico euromediterraneo, in cui si rilancia con enfasi il progetto delle autostrade del mare, quasi con uno stile da slogan pubblicitario, tralasciando che gli addetti ai lavori chiedono da tempo la realizzazione delle stesse autostrade, in modo serio, sottolineando come lo sviluppo dei trasporti nel Mediterraneo finirà per essere diretto altrove se non si investe in infrastrutture e collegamenti. Un esempio per tutti: il porto di Gioia Tauro, dotato di un importante sistema di banchine e aree di stoccaggio, ma non collegato alla rete ferroviaria. Questi investimenti, che io definisco in solitudine, credo servano davvero a poco. Nella seduta del 17 marzo 2010, la Camera dei deputati ha approvato le mozioni Lo Monte, Cicchitto, Cota ed altri concernenti misure urgenti per contrastare la crisi economica in atto. Si impegnava il Governo, tra l'altro, a valutare le opere infrastrutturali da realizzare dal punto di vista della loro sostenibilità economica ed ambientale e della loro funzionalità, concentrando le risorse verso interventi infrastrutturali realmente utili al Paese e definendo uno specifico piano infrastrutturale per il Mezzogiorno. A fronte di tali altisonanti impegni, molto poco è stato recepito poi dal Documento infrastrutture: le 28 opere pubbliche inserite dal Governo nella lista degli interventi prioritari da realizzarsi entro il 2013 non annoverano grandi novità per il Sud. Per quel che riguarda l'autostrada A3, la famosa Salerno‑Reggio Calabria, mancano 2,9 miliardi per le dieci tratte (quindi quasi 60 chilometri) che allo stato attuale non hanno nemmeno la progettazione: dalla tabella 6 risulta che sarebbero pronti i progetti di due soli di questi interventi. Tale quadro smentisce sia il Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha previsto l'ultimazione dell'intera autostrada entro il 2013, che il ministro Matteoli. Dietro cifre e percentuali che descrivono impietosamente un grave ritardo, vi sono vicende molti simili a quella della Salerno-Reggio Calabria. Basti pensare all'asse autostradale della Cisa, previsto ormai da 10 anni, del cui primo lotto è stato possibile l'avviamento solo grazie al coinvolgimento dei privati da parte della concessionaria. Non è che le cose vadano meglio nel trasporto ferroviario. Negli ultimi anni gli investimenti maggiori sono stati indirizzati all'Alta Velocità, ma a parte la linea ad Alta velocità Napoli-Bari, destinata a collegare le due grandi aree metropolitane del Meridione, il Mezzogiorno resterà sostanzialmente escluso. Il costo della tratta Napoli-Bari è di 3,2 miliardi, ma non vi è nel documento - questo è grave - alcuna indicazione di quali somme saranno effettivamente erogate e, soprattutto, quando verranno erogate. A dimostrazione di quanto il sistema ferroviario sia praticamente sottosviluppato al Sud, basta fare due esempi. Matera, innanzitutto, è l'unico capoluogo di Provincia italiano non collegato alla rete ferroviaria nazionale, dal momento che la ferrovia Ferrandina-Matera, cominciata nel 1986, non è mai stata completata. In secondo luogo, la linea ferroviaria Messina-Palermo, che corre per oltre la metà dei suoi 224 chilometri a binario unico. La situazione non è certo migliore al Centro-Nord, dove, solo per fare un esempio, l'asse ferroviario Pontremolese è un'infrastruttura prevista più o meno da vent'anni, ma non è stata ancora realizzata. Vi sono poi un paio di questioni su cui ci piacerebbe avere dei chiarimenti. Sarebbe opportuno conoscere, ad esempio, i dati precisi relativamente al coinvolgimento dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche, visto che è stato più volte dichiarato che l'ingresso di tali capitali, ai fini del finanziamento delle opere pubbliche, avrebbe contribuito a risolvere i problemi infrastrutturali del nostro Paese. Sarebbe altrettanto interessante sapere qualcosa in più sui 4,4 miliardi che il Governo conta di ricavare dai pedaggi stradali, considerato che i rappresentanti dell'ANAS hanno invece stimato l'entrata in 300 milioni di euro. Qualche giorno fa la Commissione europea ha additato l'Italia come esempio negativo di Paese che ha rinviato le riforme e si trova ora a gestire un'eredità della crisi economica più grave rispetto a chi ha agito invece per tempo. In questa particolare situazione economica, gli investimenti legati alle infrastrutture immateriali, come la banda larga - mi riferisco al settore della comunicazione - potrebbero sicuramente dare all'azione di governo un volano nell'affrontare la situazione di crisi. Al riguardo, voglio soffermarmi su una riforma importante che andrebbe fatta al più presto. La Commissione europea ha affidato agli Stati membri la libera scelta di provvedere o meno alla connettività universale. qual è la conseguenza? La divisione dei cittadini europei in due categorie: quelli di «serie A», cui la banda larga sarà assicurata a spese del proprio Stato, e quelli di «serie B», ai quali sarà negata perché lo Stato non potrà pagargliela. Non possiamo trarre - ahimè - segni incoraggianti dai documenti del Governo, che ha scelto una posizione di sostanziale immobilismo. La lista di ciò che il Governo non ha fatto conta più omissioni che azioni: ha congelato sul tavolo del CIPE gli 800 milioni di euro destinati ad investimenti nella rete; non ha investito nell'alfabetizzazione informatica; non ha previsto regole incentivanti per gli investimenti degli operatori di telefonia mobile nella banda; non ha ridisegnato un modello unitario di intervento per compensare il divario digitale; ha sostenuto un piano di riparto delle frequenze digitali che tiene fuori gli operatori del mobile. Non è una bella fotografia! In un momento di difficoltà è necessario dimostrare la capacità di investire in modo razionale sul sistema delle infrastrutture, materiale e immateriale. Il Governo si ostina invece su inutili e costosissime opere, come nel caso del ponte sullo Stretto di Messina. mi rammarico di dover dire che di fronte alle sfide che è necessario affrontare in questo Paese, il Governo non solo non vi riesce, ma neppure ci prova.

intervengo a nome del Gruppo del PD sullo schema di Decisione di finanza pubblica 2011-2013 con riguardo ai risvolti afferenti il settore primario. Potrei già considerare esaurito il mio compito, dal momento che anche questa volta l'agricoltura è radicalmente ignorata. Il Gruppo del PD in 9a Commissione ha espresso, mio tramite, il proprio orientamento contrario, fondandolo su due motivazioni: di carattere più complessivo e politico, la seconda più attinente alla competenza della Commissione. Con riguardo al primo punto, il documento in questione si pone in continuità con l'ultima manovra finanziaria, contro la quale il PD ha votato in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, non condividendone l'impostazione e stigmatizzandone l'inadeguatezza. Quanto alla seconda questione, devo dire che la stessa maggioranza, per bocca del suo relatore in Commissione, pur essendo tenuta a rassegnare parere favorevole al provvedimento in discussione, non ha potuto fare a meno di evidenziare - cito testualmente - «la necessità di integrare lo schema di decisione finanziaria con indicazioni specifiche concernenti la situazione economica del comparto agroalimentare e le prospettive inerenti allo stesso». Mi pare che si tratti di una esplicita ammissione della macroscopica negligenza del Governo, che anche in tale circostanza trascura le esigenze di un intero settore, malgrado le sofferenze che da tempo fondatamente esso manifesta. Il più eloquente indice della crisi del comparto risiede nel calo del reddito agrario, che nel 2009 in Italia è stato pari al doppio di quello mediamente registrato nell'Unione europea (12,5 in Europa, 25 per cento in Italia: siamo secondi solo all'Ungheria!). Tutto ciò è ancora più grave se si analizza, pur sommariamente, il percorso di questa prima metà della legislatura: stabilizzazione delle agevolazioni contributive nelle zone svantaggiate e montane; Fondo di solidarietà per i danni alle colture provocati dalle calamità naturali; Fondo bieticolo-saccarifero; credito d'imposta per l'internalizzazione in agricoltura; agevolazioni per il gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra; sostegno all'impresa giovanile e femminile in agricoltura, solo per citare alcuni dei problemi su cui stiamo insistendo da due anni e mezzo a questa parte, dovendo ogni volta registrare da parte del Governo l'assunzione di impegni a futura memoria, puntualmente disattesi alla prima successiva occasione utile. Così ha fatto il ministro Zaia; così sta facendo il ministro Galan. Signor Presidente, sarà maggiore o minore la capacità di comunicazione e dell'annuncio di quello che non c'è? Cambia il Ministro, ma non cambia la musica, evidentemente perché questo Governo non crede all'importanza dell'agricoltura, non investe sulla qualità, non valorizza gli enti di ricerca del settore, anzi li sopprime, non comprende la valenza promozionale e le ricadute economiche che il *made in Italy* nell'agroalimentare sarebbe in grado di indurre se fosse adeguatamente sostenuto e incentivato, non preserva il territorio di cui l'agricoltura è gestore sapiente, esponendolo ad ulteriori rischi quando le campagne vengono abbandonate perché gli imprenditori agricoli gettano la spugna. A tutto questo il Gruppo del PD si oppone, si oppone, con la consapevolezza della necessità di dare centralità all'agricoltura. Non occorrono oggi interventi episodici (peraltro mancano, come ho detto, anche quelli) anche quelli) e disconnessi da un più organico e razionale disegno. È il tempo di una vera politica agricola nazionale. Ed è anche necessario presentare il Paese con autorevolezza e con una visione nitida rispetto agli obiettivi da cogliere in sede europea, dove è imminente il negoziato sulla riforma della Politica agricola comune Il disegno, la visione, la politica mancano nell'iniziativa del Governo, e di certo il provvedimento in esame ce ne dà ulteriore conferma, il che induce a ritenere che anche per la prossima legge finanziaria le problematiche enumerate non troveranno risposta e quella opzione su una vera politica agricola nazionale non prenderà forma. Respiro corto, mancanza di strategia, tagli alle risorse e alla ricerca hanno finora caratterizzato l'azione dell'Esecutivo nei settori dell'agricoltura e della pesca, come nel comparto zootecnico, con qualche eccezione che non è lodevole, ma anzi deplorevole. Alludo alla manovra economico-finanziaria di luglio e all'inqualificabile emendamento sulle quote latte che, in barba ai vincoli dell'Unione europea, ha introdotto meccanismi premiali per chi ha operato nell'illegalità. A me pare che questo Governo sia ben lontano da quegli obiettivi alti cui puntano il Partito Democratico e i suoi Gruppi parlamentari al Senato e alla Camera, ritenendo che la competitività e il rilancio dell'economia passino anche attraverso una politica agricola matura e seria.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Vice Ministro, è la prima volta che quest'Aula discute la Decisione di finanza pubblica introdotta dalla legge di riforma della contabilità (la legge n. 196 del 2009), originata proprio da un'iniziativa della Commissione bilancio di questa Camera. È la prima volta pertanto che il Parlamento passa decisamente da una fase di mera analisi di prospettiva, quale era il vecchio DPEF, a una fase più cogente ed impegnativa, che parte sempre da un'analitica verifica macroeconomica, ma che giunge a formulare valutazioni e proposte di più aderente e concreto significato strategico e programmatico. È la prima volta della Decisione di finanza pubblica, ma non possiamo certamente scoprire oggi il tema della cessione di potere frutto della nostra partecipazione all'Unione europea, dunque dei vincoli che la partecipazione dell'Italia all'Unione europea impone anche dal punto di vista della finanza pubblica. Onorevoli colleghi, di recente, a seguito di un terribile fatto di sangue accaduto nel nostro Paese, abbiamo potuto appurare quanto siano abili molti psicologi, criminologi e investigatori ad individuare le patologie psichiatriche di un omicida immediatamente dopo che questi decide di autoaccusarsi, salvo di non saper cavare un ragno dal buco fino a quando qualcuno non confessa. Ebbene, con la DFP in un certo senso accade la stessa cosa: tanti ne criticano il contenuto, tanti sono pronti a contestarne le analisi e le prospettive, a discuterne animatamente, come già accaduto per il DPEF dell'anno scorso, ma pochi, o forse nessuno, di tali critici sono riusciti a prevedere il fatto che il nostro Paese, rispetto ad altri dell'area euro, è stato capace di non sganciarsi dal treno comunitario; anzi, è riuscito a contenere e fronteggiare la crisi economica globale e ad avviare la regolarizzazione dei conti pubblici. Tutto ciò senza avere mai pensato di aumentare la pressione fiscale a carico degli italiani, senza avere mai introdotto o aumentato alcuna tassa, senza aver fatto ricorso alle tradizionali e ben note tecniche di riequilibrio di bilancio, più prossime al concetto di bancarotta che non a quello di che non a quello di corretta contabilità pubblica. Nonostante i numerosi «corvi» della politica e dell'economia, il nostro Paese ha ripreso a crescere e a resistere. Il documento in esame oggi presenta infatti una

In base ai comunicati dell'ISTAT, nei primi due trimestri del 2010 il PIL è tornato a crescere: nel primo trimestre è aumentato dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente, e nel secondo trimestre è aumentato dello 0,5 per cento. Un dato tuttavia inferiore alla media europea, che è pari all'1 per cento, in quanto fortemente influenzato dalla crescita nettamente maggiore della Germania (2,2 per cento), ma sostanzialmente simile a quello francese e nettamente migliore di quello spagnolo. La situazione descritta nella Decisione di finanza pubblica non ci autorizza ad essere esageratamente ottimisti, ma neanche pessimisti. La situazione descritta nella DFP ci deve indurre a tenere un atteggiamento realista e costruttivo, oltre che positivo, anche perché gli strumenti che il Governo intende mettere in campo in questa fase appaiono adeguati, anche se suscettibili di ulteriori implementazioni, anche frutto di questo dibattito. Una implementazione funzionale è connessa alle politiche riformatrici riguardanti la giustizia e i suoi tempi biblici. Altre potrebbero essere la scuola, il lavoro, le procedure burocratiche, la gestione e la razionalizzazione delle opere pubbliche, la sanità, di cui di cui si parla in questi giorni purtroppo per le vittime che ha prodotto. Insomma, le varie riforme che sono state annunciate possono certamente determinare economie di scala di scala e altresì risorse destinabili a nuove politiche di sviluppo e di sostegno alla produzione, al lavoro, alla famiglia, migliorando certamente la situazione, anche in virtù delle indicazioni, dei suggerimenti e delle politiche comunitarie. Analoghi risultati virtuosi sono inoltre non solo auspicabili ma anche ipotizzabili con la messa a regime del federalismo fiscale, e in particolare del provvedimento del Governo sui costi e sui fabbisogni standard di Comuni e Province. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia recentemente ha affermato che nessuno sviluppo è ipotizzabile se i conti dello Stato non sono a posto. Aggiungo a questo concetto che condivido quale i conti dello Stato vanno a posto più rapidamente se l'economia cresce con maggiore velocità e l'occupazione aumenta di pari passo. Comprendo che questa può apparire una affermazione lapalissiana, ma forse proprio per questo va ben spiegata: intendo dire che il superamento della crisi è certamente supportato dalle politiche pubbliche messe in campo dal Governo e più in generale dalla politica, ma non può fare a meno né di una diversa e più dinamica organizzazione del lavoro, né di un rinnovato entusiasmo dell'imprenditoria, né di una armonica perequazione infrastrutturale del Paese. bisogna dire con chiarezza, onorevoli colleghi, che la ripresa descritta e programmata nella Decisione di finanza pubblica, per sortire i virtuosi effetti ipotizzati, non può essere negativamente influenzata né da una Confindustria che invece di guardare allo sviluppo economico del Paese guarda al prossimo Governo, né da una parte del sindacato che come modello industriale, guarda ancora ai *soviet* e alla loro organizzazione, già sconfitta dalla storia, piuttosto che alle nuove tecnologie; ma soprattutto, non può essere negativamente influenzata neanche da una crescita infrastrutturale sperequata nel Paese. Nella relazione sul programma delle infrastrutture strategiche allegato allo schema di DFP si indica un dato estremamente interessante riferito agli investimenti per il Sud, che passano dall'8-10 per cento della media del passato cento: dato che conferma le colpe dei precedenti Governi. Certo, l'inversione di tendenza è significativa e importante, ma se al Sud si investirà solo un terzo delle somme disponibili e altrettanto al Centro e al Nord, si sta ipotizzando solamente il mantenimento dell'attuale condizione sperequata. Una condizione che supera di gran lunga il netto abbandono del passato, ma che, allo stato, rende forse esageratamente lenta quella perequazione infrastrutturale di cui il Paese ha bisogno, sia per marciare alla stessa velocità in ogni sua area geografica, sia per rendere pienamente operativo il federalismo fiscale che - lo fiscale che - lo sottolineo - si fonda proprio sulla perequazione infrastrutturale e sull'armoniosa crescita del Paese nel suo complesso. Questo è un dato che penso questo Parlamento e il Governo debbano sempre avere ben chiaro: il federalismo si realizza attraverso e previa la perequazione infrastrutturale. c'è, esiste, ma adesso bisogna pensare ai dettagli, perché sono proprio i dettagli che rendono nitida l'immagine del risanamento risanamento e nitido il progetto di sviluppo che il Paese intende realizzare, che il Governo sta realizzando e che la politica, sia pure tra mille difficoltà, non può che assecondare, per renderlo più celere ed efficace.

cui si chiede al Ministro dell'interno di riferire in merito ad una difficilissima e incresciosa situazione relativa al Comune di Cercola, in provincia di Napoli, che conta circa 20.000 abitanti. Nell'interrogazione è documentata una serie di atti gravi, di patenti illeciti amministrativi e contabili, fatti accertati, oltre che di evidenti contiguità con persone inquisite o arrestate. Un Comune che era sostanzialmente sano, con un bilancio florido fino al 2009, è oggi veramente compromesso da molti punti di vista. Chiediamo al Ministro dell'interno se non ritenga